Comunico, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, che la delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa è convocata domani, 13 aprile 2023, alle ore 9, presso la Camera dei deputati, Palazzo del Seminario, quarto piano, Auletta delle delegazioni, per procedere alla propria costituzione.

per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" (564)

è un problema annoso, che i senatori vorrebbero che le riformulazioni da parte dei Ministeri arrivassero con tempi più celeri, ma purtroppo questa è la prassi e ne dobbiamo prendere atto.

reca una modifica all'articolo 2, comma 3, della legge 23 marzo 2023, n. 33, recante deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), prevedendo tra l'altro che allo stesso competa l'adozione con scadenza triennale e aggiornamento annuale, previa intesa in sede di Conferenza unificata, del Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana e del Piano nazionale per l'assistenza e la cura delle fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana. Il comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione proroga i termini per l'esercizio della delega per la riforma dei criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, le revisioni del numero degli incarichi semidirettivi, la revisione dei criteri di accesso alle funzioni di legittimità, del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative e degli uffici giudicanti e il riordino della disciplina del collocamento in posizioni di fuori ruolo dei magistrati ordinari amministrativi e contabili, conferita al Governo con la legge n. 71 del 2022. Per quanto riguarda il decreto-legge, si illustra di seguito una sintesi dei contenuti, evidenziando le modifiche approvate in sede referente. I commi da 1 a 3 dell'articolo 1 prevedono che i regolamenti di organizzazione dei Ministeri possano procedere alla riorganizzazione della struttura di livello dirigenziale generale ovvero dell'unità di missione di livello dirigenziale generale preposta al coordinamento delle unità di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR e a quelle delle amministrazioni centrali. Tengo a sottolineare che, durante le audizioni, praticamente la quasi totalità degli auditi è stata favorevole a questo provvedimento di *governance*.

n. 108, in materia di *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza. In particolare, è soppresso il tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, così come ogni riferimento normativo a tale organo. Le funzioni di coordinamento e cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale sono trasferiti alla cabina di regia per il PNRR, alle cui sedute, specificamente dedicate, partecipano anche i rappresentanti degli enti e delle organizzazioni che finora avevano costituito il tavolo permanente. Sono introdotte infine alcune modifiche relative ai compiti e alle funzioni della Segreteria tecnica istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di supporto alle attività della cabina di regia.

modifica talune disposizioni riguardanti il monitoraggio e la rendicontazione del PNRR, specie sostituendo - presso il MEF-RGS il Servizio centrale per il PNRR con l'ispettorato generale per il PNRR, nonché istituendo presso il medesimo Ministero due posti di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca. La lettera *f)* novella alcune disposizioni riguardanti il controllo e l'audit del PNRR, specie autorizzando la stipula di convenzioni con pubbliche amministrazioni per la realizzazione del programma di valutazione in itinere ed *ex post* del PNRR, aumentando il numero degli incarichi di livello dirigenziale non generale, consentendo la stipula di protocolli di intesa con la Guardia di Finanza anche alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, agli enti locali e agli altri soggetti pubblici che provvedono alla realizzazione degli interventi del PNRR al fine di rafforzare le attività di controllo, nonché prevedendo per la RGS la possibilità di promuovere misure finalizzate alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure di controllo del PNRR al fine di assicurare il coordinamento dei controlli e di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei soggetti attuatori. La lettera *f-bis)*, introdotta in sede referente, novella - a fini di coordinamento - la medesima disciplina della Governance relativamente al coordinamento della fase attuativa del PNRR. L'articolo 1, dispone il trasferimento delle competenze regolatorie sui servizi pubblici locali non a rete dalla Presidenza del Consiglio al Ministero delle imprese e del *made in Italy*. L'articolo 2 istituisce - fino al 31 dicembre 2026 - una Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio, disciplinandone funzioni e composizione.

mia volta un ringraziamento alla Commissione bilancio, al suo Presidente e a tutti i colleghi per il lavoro svolto, nonché al Ministro e al Sottosegretario. Abbiamo esaminato un decreto complesso e delicato, come quello in discussione, approfondendo nel merito molte questioni e rispettandone sempre l'obiettivo principale che - lo ricordiamo - è quello di assicurare la tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, attraverso il rafforzamento della capacità amministrativa e la semplificazione dei vari In questa prospettiva, è stato molto importante il contributo delle audizioni preliminari, che hanno valorizzato il dibattito in Commissione con istanze e proposte che sono state tradotte tradotte in emendamenti dai Gruppi parlamentari. La trattazione del provvedimento è stata quindi costruttiva e ci consegna un testo arricchito sotto numerosi aspetti, che rimettiamo all'esame dell'Assemblea. In maniera concisa e senza pretesa di esaustività, vorrei riepilogare con il mio intervento alcune misure previste dall'articolato, concentrandomi in particolare su quelle di recente introduzione, inserite nel corso dell'esame in sede referente. La struttura del decreto-legge - lo rammento - si articola in tre parti, suddivise a loro volta in titoli e capi. La prima parte contiene disposizioni volte alla riorganizzazione della della *governance* per il PNRR; lo scopo è quello di rafforzare il sistema di coordinamento, gestione, attuazione e monitoraggio delineato dal decreto-legge n. 77 del 2021, anche alla luce dell'istituzione dell'autorità politica delegata in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza. La seconda parte reca disposizioni atte a rafforzare la capacità amministrativa e a snellire le procedure. La terza parte reca disposizioni in materia di politiche di coesione e di politica agricola comune, nonché di politiche giovanili. Rispetto al testo originario del decreto-legge, le novità principali che mi accingo a illustrare riguardano: la semplificazione delle procedure di accesso da parte delle stazioni appaltanti alle risorse dei fondi per il riconoscimento della revisione dei prezzi; l'emendamento che rende che rende più agevole, per gli enti locali, il ricorso ai contratti di somministrazione di lavoro per far fronte alle attività del Piano nazionale di ripresa e resilienza; la risoluzione della problematica Pinqua (Programma innovativo nazionale sulla qualità dell'abitare) mediante la destinazione di risorse aggiuntive, per cento dell'importo già assegnato, per gli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e oggetto di procedure di affidamento e di accordi quadro; il riconoscimento dell'anticipazione di ulteriori risorse per il piano banda ultralarga; le semplificazioni per l'affidamento dei progetti connessi alla realizzazione delle opere per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica del 2025; la nomina di un Commissario straordinario per accelerare la realizzazione degli interventi occorrenti per lo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026; la nomina di un commissario straordinario al fine di garantire la realizzazione della linea 2 della metropolitana della città di Torino; l'emendamento che prevede il coinvolgimento del GSE nell'attuazione degli interventi di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; le semplificazioni per l'installazione di infrastrutture per la produzione di energia *green*; gli emendamenti che estendono la stabilizzazione anche al personale assunto per le esigenze del Piano nazionale di ripresa e resilienza da parte di Regioni, Province, Città metropolitane ed enti locali. Inoltre, con riguardo alle politiche di coesione, segnalo la norma che consente l'utilizzo delle risorse cosiddette liberate, ovvero le risorse che derivano dalla rendicontazione sui programmi europei, nazionali e regionali di spese già sostenute con fondi pubblici derivanti dal bilancio statale. Importante, sempre con riferimento alle politiche di coesione, è anche la messa in sicurezza della falda da realizzare nel sito di Piombino, nelle aree della società Aferpi SpA.

soffermarmi sul metodo, dando atto al Governo e, in questo caso, al ministro Fitto e ai Sottosegretari, di aver portato avanti un dialogo costruttivo con le opposizioni. Per questo devo anche ringraziare il presidente della Commissione bilancio Calandrini, perché aver preso il tempo giusto, necessario per analizzare il provvedimento e gli emendamenti, in un dialogo costruttivo con l'opposizione, credo faccia bene al Paese. In questo caso, infatti, non stiamo semplicemente ponendo le condizioni perché si spendano delle risorse, ma ci stiamo giocando la credibilità del Paese nel contesto europeo e internazionale. Prima di entrare nel dettaglio dei singoli emendamenti, vorrei soffermarmi su questo punto, che per me è essenzialmente politico: troppe volte, quando parliamo del PNRR, ci concentriamo sulla capacità di spesa e diciamo che il nostro Paese ha problemi strutturali nell'incapacità di spendere le risorse che vengono dall'Europa. Questo è sicuramente vero, ma occorre fare attenzione a non cadere nell'errore di pensare che il PNRR si riduca a un tema di spesa, perché ciò che è davvero centrale è quali delle risorse che oggi mettiamo in campo saranno capaci di creare crescita e investimenti.

Se l'Europa ci dà queste risorse è perché la condizione per poterle utilizzare è finalizzata a realizzare riforme che da troppi anni non riusciamo a fare. Ecco perché in Assemblea interveniamo quando c'è il tema della concorrenza, non piegandoci alle singole richieste delle corporazioni. Ecco perché, signor Presidente e signor Ministro, chiediamo che dalla capacità di spendere le risorse del PNRR passino il futuro, la crescita e la capacità di investire in infrastrutture importanti per il nostro Paese. Questo è essenzialmente un tema politico e riguarda come ci si rapporta al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il quale, come ricordo sempre, si chiama per un certo motivo Next generation EU, ovvero perché dev'essere fatto nella consapevolezza che andiamo a prendere le risorse a debito per le future generazioni *(Applausi)* ed è per loro che dobbiamo spendere questi soldi, quando parliamo infrastrutture e di transizione ecologica e digitale. dei punti e dei singoli emendamenti che sono stati approvati e che per il Gruppo Azione-Italia Viva-RenewEurope sono importanti. C'è il tema di Italia sicura, sul quale sapete che abbiamo fatto una battaglia. anche che l'emendamento non ci soddisfa appieno, perché poniamo un tema di trasversalità della Protezione civile, nella necessità che rientri sotto la Presidenza del Consiglio dei ministri. Prendiamo atto che c'è la volontà di

noi ci giochiamo davvero molto, piuttosto che dover intervenire sempre inseguendo la dittatura dell'emergenza di crisi e di eventi che purtroppo tempestano strutturalmente il nostro Paese. Un altro elemento, signori

in esame dev'essere letto in maniera integrata con il prossimo decreto-legge, che è quello su REPowerEU, e ci sembra giusto non forzare la mano sul tema del PNRR per

riusciremo a utilizzarle non solo perché le spenderemo in senso opportuno, ma perché realizzeremo le infrastrutture che ci consentiranno di fare un

primo riguarda il tema dei ricercatori e voi sapete quanto sia importante per un mondo della ricerca che ci guarda e che chiede esattamente, attraverso il PNRR, che sia possibile fare un passaggio tra il mondo della ricerca e il mondo dell'impresa,

che chi oggi ha un contratto come ricercatore a tempo definito possa lavorare nel mondo delle imprese. Noi dobbiamo sempre creare questo collegamento tra il sapere e il saper fare, nonché tra l'università e il mondo imprenditoriale, perché questa è una riforma importante per il Paese. Un altro emendamento molto significativo e molto rilevante per noi è quello che riguarda l'utilizzo delle risorse del PNRR per l'edilizia residenziale universitaria. Voi sapete quanto sia difficile oggi per uno studente fuori sede trovare un alloggio nelle città che ospitano le università italiane. Noi sappiamo che il PNRR mette a disposizione delle risorse, ma sappiamo che fino ad oggi la licenza per poter fare queste residenze era una licenza residuale,

Arrivo così a un punto per noi importante. Come dicevo già nell'audizione del ministro Fitto, noi consideriamo che aver agganciato il tema della scadenza del PNRR a quello della scadenza dei fondi di coesione sia una scelta strategica importante. auspicheremmo maggiore chiarezza sul modo in cui i progetti possono transitare da una linea di fondo all'altra, ma sono sicuro che su questo state immaginando un percorso in cui la scelta non verrà fatta sulla base della scadenza temporale, ma della priorità

il Governo si assume la responsabilità di intervenire sulla *governance*, nell'idea che la sua semplificazione possa portare a mettere a terra questi progetti.

il Governo si assume la responsabilità di togliere l'alibi che la *governance* non fosse funzionale a realizzare i progetti e a spendere queste risorse nella via delle riforme. membri del Governo, vi valuteremo alla prova dei fatti, sapendo che dalla nostra parte ci saranno sempre proposte migliorative, tese a realizzare non solo la capacità di spesa dei progetti, ma le riforme che l'Europa ci chiede e che a noi servono da troppo tempo. il decreto-legge al nostro esame rappresenta una sorta di tagliando alla macchina che si occupa del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Credo che siamo tutti convinti che l'interesse dell'Italia sia di ricominciare a crescere a un ritmo sostenuto e intraprendere un percorso virtuoso tra le grandi potenze economiche. Le risorse del PNRR possono certamente aiutare sulla strada della crescita economica e a raggiungere nuovi livelli di produttività. Sarà altresì fondamentale ultimare il percorso di riforme legate alla piena attuazione del Piano. Credo che attuare tutte le riforme che possono rendere il Paese più competitivo debba essere il nostro obiettivo prioritario. Ecco perché questo decreto è importante: si interviene, migliorandolo, sul sistema della *governance* del Piano e sulle regole per rafforzare la capacità amministrativa dei soggetti che devono attuare gli interventi previsti dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, accelerando e semplificando le procedure. in discussione interviene anche su diverse disposizioni per l'attuazione delle politiche di coesione, delle politiche agricole e delle politiche giovanili. È un testo che contiene diverse disposizioni volute anche dai ministri di Forza Italia Alberti Casellati, Bernini, Pichetto Fratin e Zangrillo, che si trovano a dare attuazione al Piano per le parti di loro competenza. È un testo arricchito anche del lavoro del Gruppo Forza Italia, che ha presentato ulteriori proposte migliorative, accolte dalla Commissione bilancio del Senato, che nascono dalle esigenze dei territori e dalle categorie produttive. Mi sembra che l'importanza del successo dell'attuazione del Piano sia stata ribadita un po' da tutti i Gruppi parlamentari, non solo di maggioranza, ma anche di opposizione, che hanno visto approvate molte delle loro proposte emendative. Si è capito cioè che attuare riforme strutturali il più condivise possibile e dare piena attuazione al Piano significa contribuire alla modernizzazione del Paese. Insomma, non è solo questione delle risorse che possono aiutare la crescita del PIL in questi anni fino al 2026, ma si tratta di porre le basi per un'Italia che corra a una velocità maggiore di quella a cui sta marciando adesso. Certamente, meglio si spende e meglio è. Lo scopo del decreto-legge in discussione è anche questo: migliorare i meccanismi di *governance* complessiva del Piano; migliorare i controlli e ottimizzare i risultati, anch'essi legati alla spesa. Soprattutto, però, ci si è posti l'obiettivo di semplificare le procedure che renderebbero di difficile attuazione alcune parti del Piano. Non ci sono quindi ritardi, ma la messa in funzione di una macchina complessa, il cui controllo viene centralizzato e le cui strutture periferiche vengono messe nelle condizioni di operare. Inoltre, la nuova responsabilizzazione della struttura centrale, di quella ministeriale e di quelle che danno pratica attuazione alle misure del Piano le mette nella condizione di operare al meglio. È fondamentale anche aver messo in questo campo, in caso d'inerzia o ritardo di un'amministrazione, i poteri sostitutivi in caso di mancato rispetto da parte delle Regioni degli impegni finalizzati all'attuazione del PNRR. Questo prevede il ruolo del commissario che s'incarica dell'esecuzione dei progetti PNRR o PNC, assicurando il coordinamento operativo delle varie amministrazioni e dei diversi soggetti coinvolti. Per quanto riguarda le infrastrutture, che, come sappiamo, scontano il rincaro delle materie prime e dei materiali del settore delle costruzioni, al commissario vengono affidati i poteri che sono in capo al commissario straordinario delle grandi opere. Lo stesso Governo dimostra di credere nella realizzazione del Piano, tanto che in caso di dissenso, diniego e opposizione alla realizzazione di un intervento previsto dal PNRR, si prende le proprie responsabilità. Viene infatti attribuito il potere d'impulso per rimettere la decisione al Consiglio dei ministri anche al Ministro competente, oltre che alla struttura di missione del PNRR. tempo, vengono introdotte nuove norme volte a favorire da parte del Ministero dell'economia e delle finanze il controllo e il monitoraggio della spesa degli interventi legati sia al PNC sia al PNRR. Adottare per le nuove opere da realizzare le procedure già previste per l'edilizia penitenziaria, ferroviaria e giudiziaria, in materia di conferenze dei servizi, di valutazioni di impatto ambientale e acquisizione degli assensi dei beni culturali, potrebbe essere un vero punto di svolta. Ci sembra un importante passo in avanti anche la previsione che il demanio e il Ministero della difesa possano mettere a disposizione i loro immobili dismessi per realizzare alloggi universitari, infrastrutture sportive ed energetiche da fonti rinnovabili. un decreto che segna una serie di semplificazioni per attuare un piano ambizioso, ma largamente realizzabile. Ci auguriamo che determinate procedure, ora velocizzate, aprano la strada per un cambio di paradigma, cioè un nuovo rapporto tra lo Stato e chi lavora per realizzare le opere di cui il settore pubblico è committente. È il modo migliore per far ripartire il Paese, assieme alle tante semplificazioni amministrative previste, volute dal ministro Zangrillo, a cui va il nostro plauso. L'augurio è proprio quello che si segni un nuovo rapporto tra Stato e gestione delle risorse pubbliche, tra Stato e cittadino, che aiuti il Paese a fare quel cambio di velocità verso la modernizzazione che tutti auspichiamo e che adesso vediamo più facile da raggiungere.

credevo oggi di intervenire su un provvedimento in materia di semplificazione, ma evidentemente mi sbagliavo, perché qui, piuttosto che semplificarsi, la questione si complica. Si getta sul Piano nazionale di ripresa e resilienza un velo che in maniera irreversibile ne rallenterà l'attuazione, pur essendo il più importante piano che l'Italia abbia mai potuto vedere. In campagna elettorale, come noto,

signori del Governo, io credo che sia arrivato effettivamente il momento di dire a quest'Assemblea e al Paese intero per cosa ritenevate effettivamente di essere pronti. Mi permetto di porgervi una piccola domanda: lo direste ancora? L'umiltà di certo non è un tratto distintivo di questa maggioranza, ma qui vi si chiede di essere onesti e corretti nei confronti del presente e del futuro di un Paese che chiede risposte; onesti e corretti nei confronti di tutti e di chi vi ha scelto perché ha creduto a quel «siamo pronti». Il punto però è proprio questo. Quando in quest'Aula e nelle piazze c'era da urlare il vostro dissenso, lo avete fatto benissimo, con la ben nota *verve* politica che ha caratterizzato il vostro modo di fare e di intendere l'opposizione. Ora che siete dall'altra parte, il tono necessariamente è cambiato e vi ritrovate a sussurrare e a farfugliare soluzioni improvvisate che mancano di visione programmatica e strategica. Chi vi osserva capisce lo stato di costante e preoccupante confusione, che è la chiave di lettura di quella che vi piace definire come la vostra rivoluzionaria agenda politica. Abbiamo visto abbastanza? Io purtroppo credo di no e vado al merito del provvedimento. Partiamo dalla questione della *governance*, che viene completamente smantellata per essere accentrata a Palazzo Chigi. è il momento giusto per far decadere tutte le strutture tecniche tirate su nei Ministeri perché...». La questione non è chiara. Forse solo perché dovete mettere la vostra bandiera di destra sull'attuazione del piano, senza considerare minimamente che garantire la continuità su programmazione e monitoraggio è una questione di buonsenso che va ben oltre la vostra bandierina; senza considerare che la *governance* è una questione meramente tecnica e non politica; senza considerare che i soldi faticosamente ottenuti durante l'emergenza pandemica non sono né di destra, né di sinistra, ma sono degli italiani. Avete detto che il cambio di *governance* si è reso necessario a seguito dell'esperienza acquisita nel contesto del PNRR; quindi, invece di correggere il tiro, decidete di sterzare violentemente, senza considerare tutti gli effettivi ritardi

asincrone, ad esempio, anche con il codice degli appalti. Infatti, per semplificare gli interventi di edilizia scolastica avete deciso di muovervi in deroga alle normative già previste per l'aggiudicazione dei contratti sotto soglia mediante l'affidamento diretto di servizi e forniture

ve lo abbiamo detto tutti, anche fuori dal Parlamento, ma niente, vi siete innamorati e intestarditi sul cosiddetto modello Genova, a dispetto della maggior tutela e trasparenza degli affidamenti e della qualità della progettazione che, in un ambito così sensibile e delicato qual è proprio quello dell'edilizia scolastica, appare ancora più rilevante. Troppo spesso i partiti di centrodestra hanno invocato il modello Genova come la panacea di tutti i mali legati alla lentezza nell'attuazione dei contratti pubblici del nostro Paese. In maniera miope non siete mai riusciti a comprendere il caso, l'*unicum* delle procedure previste per la ricostruzione del ponte Morandi di Genova, che non potranno mai diventare parametro ordinario utile a colmare il *deficit* cronico rappresentato dalla capacità di progettazione della pubblica amministrazione. In ambito infrastrutturale avete deciso di tagliare sulle normative previste dal codice dell'ambiente; avete deciso di tagliare sulle conferenze unificate, sulle conferenze Stato-Regioni, optando per il silenzio-assenso. Avete deciso di non ascoltare nessuno, ma del resto non è una novità: diciamo che questa è una delle tante caratteristiche e peculiarità dell'attuale Esecutivo. Ebbene, voi avete il diritto di non ascoltare nessuno, esattamente come noi abbiamo il il dovere di ricordarvi che le imprese italiane vedono nel loro orizzonte un'opportunità legata ai bandi di gara, ma, al contempo, percepiscono le difficoltà legate alla forte contrazione da parte degli istituti bancari della concessione delle garanzie fideiussorie necessarie all'accesso ai bandi pubblici. Siamo qui dunque

C'eravate voi allora e ci sarete anche dopo, prossimamente, quando vi accorgerete di aver nuovamente sottovalutato questo aspetto, l'odioso fenomeno dei bandi di gara andati deserti, che non può essere sconfitto dall'unica soluzione che siete riusciti che siete riusciti a individuare, ovvero l'affidamento diretto, al posto della massima partecipazione delle imprese e della trasparenza. Abbiamo tentato di aiutarvi con proposte ed emendamenti, ma voi avete deciso di tirare dritto per la vostra strada, con quella spocchia e arroganza che ormai contraddistinguono questo Esecutivo, perché - possiamo dircelo - state creando scompiglio e incertezza nei mercati; siete il Governo della retromarcia, senza visione sistemica del Paese, che punta solo a piazzare le proprie bandierine. Avete deciso di assumervi questa responsabilità; ne avete la legittimità, ma, ancora una volta, non sarete voi a pagare per queste vostre scelte. A pagare saranno i cittadini e le imprese che in questo grande Piano Marshall denominato PNRR hanno riposto grande speranza, ahimè invano, purtroppo. Siamo pronti, dicevate. Colleghi della maggioranza, membri del Governo, lo dico con sincero dispiacere: ci avete stupiti. Non ci aspettavamo tanta incompetenza e tanta improvvisazione; siamo noi che non eravamo pronti! Il Paese non era pronto allo spettacolo che state mettendo in scena. Ad oggi la vostra abilità più evidente è quella di essere riusciti ad andare oltre ogni spiacevole aspettativa. *(Applausi)*. di urlare, e lo dicevo poc'anzi, ma c'è bisogno che qualcuno di voi torni a farlo, quantomeno per provare a svegliare tutti gli altri. Noi ci stiamo provando in tutti i modi, ma forse avete bisogno di sentire una voce amica: svegliatevi e aprite gli occhi sul Paese! Un Paese che non può permettersi il lusso di dormire, e che, anzi, avrebbe il diritto di trasformare in realtà il sogno di un futuro più giusto per i propri figli, sfruttando nel migliore dei modi la grande opportunità che ci è data dai fondi ottenuti da Giuseppe Conte e dal suo Governo. Certo, dite voi, restituiamo i fondi del PNRR che sono troppi e difficili da gestire e giochiamoci la carta del ponte sullo Stretto: dirlo non costa nulla, è una buona propaganda effettivamente; ma da quanti anni se ne parla? È così urgente o forse è il solito *spot* di un Ministro che ormai ha detto tutto e il contrario di tutto, essendo anche stato contrarissimo al ponte, come qualcuno ricorderà come me. Signor Presidente, mi permetto di concludere questo intervento con un suggerimento all'Esecutivo guidato dalla signora Meloni. Il primo ponte che dovreste impegnarvi a costruire è quello tra voi e il Paese reale *(Applausi)*, quello tra voi e la gente

Voi al posto nostro avreste continuato a urlare, ne sono certa, come avete sempre fatto. Noi vi tendiamo una mano: l'Italia non può permettersi di fallire, sarebbe un prezzo troppo alto per la Nazione. Spero per voi e per l'Italia che almeno di questo siate consapevoli.

Cerchiamo di fare un po' di ordine su questo PNRR. La situazione chiaramente complicata perché siamo nella fase più difficile, quella di avvio dei cantieri, e abbiamo tante risorse da spendere in poco tempo. Le risorse sono di due tipi: quelle a fondo perduto, che chiaramente vanno spese fino all'ultimo centesimo - ci mancherebbe altro! - e le risorse a prestito, che vanno spese anch'esse il più possibile, diciamo tutte e però con un surplus di responsabilità. Mi spiego. Le risorse a fondo perduto sono, appunto, a fondo perduto: è chiaro che se le usi per fare feste e fuochi d'artificio hai buttato via dei soldi, ma almeno non devi restituirle. Le risorse a prestito le devi restituire: quei 123 miliardi vanno restituiti tutti fino all'ultimo centesimo,

Ma all'epoca, almeno, i tassi erano vicini allo zero, quindi restituivi solo il capitale; adesso c'è anche un bel 3-4 per cento di interessi. Quindi, c'è un *surplus* di responsabilità. Tradotto: ogni investimento che si fa deve rendere di più del costo, altrimenti hai buttato via i quattrini. Questo è il concetto chiave - lo sa benissimo il ministro Fitto - ed è una grande responsabilità. ovvio che la maggior parte di questi investimenti - e dico giustamente investimenti - devono essere produttori di PIL.

la prima distinzione, porto la mia esperienza da ex Ministro del turismo: come siamo riusciti ad allocare tutte le risorse velocemente e in buona parte a spenderle?

Se si destina mezzo miliardo di euro, che poi sono diventati 900 milioni, a strutture ricettive per migliorarle, quelle fanno un investimento e fanno subito PIL; l'anno dopo hai il credito d'imposta, hai fatto PIL e hai speso tutte le risorse.

Quindi, due miliardi si possono spendere subito. Diverso è quando si entra nella spesa pubblica. Allora, sulla spesa pubblica la distinzione è tra grandi e piccoli interventi. Sui piccoli interventi sappiamo che c'è la difficoltà della frammentazione e la scelta è fra gli interventi che possono essere fatti e quelli che non possono essere fatti. Vuol dire tanti appalti e tanti quadri economici da rivedere in base ai prezzi. Questo è il problema soprattutto degli investimenti più piccoli, dei piccoli e medi Comuni, perché se la disponibilità è dell'80 per cento salta tutta l'opera.

Sulle grandi opere, invece, vi è la classica difficoltà italiana, causata dalla sindrome NIMBY (non nel mio giardino). Allora, faccio l'esempio degli esempi, che per un milanese è il più facile: sapete quanti anni ha il primo termovalorizzatore di Milano? Ce ne sono tre a Milano e tredici in Lombardia: il primo termovalorizzatore di Milano ha cinquantacinque anni, la mia età. A Roma si discute se, forse, farne uno. A mio avviso ne andrebbe fatto uno ogni due milioni di abitanti: fine. È un'altra cosa da fare subito, semplice. Veniamo alla conclusione: come mai questa scelta, tutta italica, di chiedere così tante risorse a prestito senza tener conto delle conseguenze, anche reputazionali? Infatti, poi, poi, rinunciare a una parte di queste risorse è una conseguenza reputazionale per il sistema Paese, ma probabilmente si è mutuato quello che si fa puntualmente col Fondo sviluppo e coesione.

non c'è problema, c'è la rimodulazione, termine burocratico che sta per rinvio. Quindi, noi strutturalmente emettiamo BOT, emettiamo debito pubblico per fare ipotetiche azioni azioni di investimento e poi rimoduliamo, cioè rinviamo e non le facciamo. Perché? Perché spesso è più importante, purtroppo, vendere le risorse portate a casa piuttosto che le risorse effettivamente spese.

Quando la politica imparerà che il titolo sul giornale si fa quando l'opera è fatta, forse sarà tardi. Grazie e buon lavoro. il Piano nazionale di ripresa e resilienza rappresenta uno strumento imprescindibile e straordinario per costruire il futuro del nostro Paese. Per questo, la discussione alla quale abbiamo assistito nelle ultime settimane ritengo sia stata totalmente inadeguata. Lo è rispetto al valore strategico del Piano e, per certi aspetti, non è neanche stata una discussione responsabile. Il Paese, dopo la pandemia e la crisi internazionale provocata dall'aggressione della Russia all'Ucraina, vive uno stato di emergenza che rischia di minare lo sviluppo e il futuro. La crisi economica colpisce le aree più deboli d'Italia. Tra i nostri territori crescono sempre di più le differenze. Sono migliaia le imprese che rischiano di chiudere facendo impennare ancora di più la disoccupazione e la desertificazione - perché di questo si tratta - di molte aree. e sono prive di senso le discussioni sulla quantità dei finanziamenti concessi dall'Europa o sulle eventuali responsabilità dei Governi precedenti. Ci troveremmo davanti a un problema reale se le risorse non ci fossero, invece l'attenzione credo debba essere concentrata esclusivamente sullo sforzo che deve essere fatto adesso per non disperdere le risorse e per riuscire a realizzare gli interventi programmati. Questo è il problema che va affrontato qui ed ora e risolto, senza cercare altri alibi e giustificazioni. Siamo preoccupati per l'emergere invece di un quadro di inadeguatezza complessiva dell'attuale Governo di centrodestra, che dopo aver accumulato ritardi sul PNRR sembra voler mettere le mani avanti per nascondere le proprie responsabilità. Del resto, le stesse divisioni interne alla maggioranza non lasciano ben sperare. Ci preoccupa e dovrebbe preoccupare tutti che la stessa presidente Meloni si sia trovata costretta a dover smentire un pezzo della sua maggioranza, cioè la Lega, che aveva addirittura immaginato la possibilità di rinunciare a questi fondi europei. questa grande confusione si debba rispondere partendo dai problemi fondamentali che ancora non hanno trovato adeguato spazio neanche nel dibattito avvenuto in Commissione bilancio. proseguire con continue riformulazioni dei progetti, modificando in modo caotico le misure del PNRR, non sembra essere una strada che possa portare a risultati concreti. Le stesse riformulazioni, del resto, come propone l'Esecutivo senza adeguati approfondimenti, rischiano solo di amplificare la confusione, dilatando l'impianto burocratico-amministrativo che già sta mettendo in difficoltà le amministrazioni locali. La sostanza della difficoltà è altrove: anche se il Governo continua a non volerne prendere atto, moltissimi dei ritardi accumulati nella programmazione derivano dall'insufficienza del personale in forza nelle pubbliche amministrazioni a tutti i livelli. Per questo abbiamo presentato degli emendamenti, uno in particolare, in Commissione, per chiedere la stabilizzazione dei lavoratori precari a seguito del superamento dei concorsi pubblici indetti dall'Agenzia territoriale di coesione. Si tratta di circa 2.000 persone. Quell'emendamento è stato riformulato, forse riusciremo ad ad approvarlo, ma non basta. È necessario affrontare la questione degli enti locali in maniera più complessiva. Come lei sa, signor Ministro, molti degli enti locali italiani sono in dissesto o in predissesto e rischiano di non poter assumere le figure professionali che servono. Questo decreto non riesce a colmare le lacune e i problemi di questi enti. Servono interventi volti a potenziare le amministrazioni pubbliche. punto, però, di essere ancora più chiaro, perché le dichiarazioni di quella discussione, di cui parlavo all'inizio, ci preoccupano, perché, per eventuali amministrazioni in difficoltà, non si possono né si devono prevedere interventi punitivi e pericolosi per la stessa unità nazionale. Sono urgenti, invece, interventi di sostegno, magari anche prevedendo un sistema di aiuto per rendere uniformi gli *standard* di *governance* delle risorse in tutto il Paese. Esattamente il contrario delle proposte estemporanee arrivate da diversi esponenti del centrodestra, che vorrebbero applicare il principio di dirottare le risorse non spese alle amministrazioni in grado di spenderle. Ministro, credo che lei comprenda la gravità di questa affermazione che un pezzo della maggioranza ha cristallizzato negli scorsi giorni. prima si aggrava la crisi degli enti locali più deboli, soprattutto nel Mezzogiorno e ora si vorrebbero spostare le risorse. Siamo all'ennesima trovata per sviare il dibattito pubblico dai problemi reali e per continuare ad aumentare il divario fra le aree più ricche del Paese e quelle più fragili. Altra questione che dovrebbe essere affrontata in maniera urgente è quella dell'aumento dei costi dell'energia e delle materie prime, per l'impatto che tali aumenti hanno sulla spesa e sulla gestione del PNRR. Sono costi che aggravano le difficoltà per le amministrazioni comunali, che non riescono nemmeno a pagare le bollette. tali aumenti dei costi di energia e materie prime possano determinare un costo, nei cantieri del PNRR, di oltre il 20 per cento. Dovremmo, dunque, discutere di come utilizzare almeno parte delle risorse disponibili per coprire questi aumenti. Altrimenti, ci troveremo a dover fare i conti con una lunga serie di progetti incompleti. Io spero che il Governo sappia che questo decreto-legge non riesce nemmeno a dare una risposta alle criticità delle università. Le università hanno il compito di gestire la missione 4. Nell'ambito del PNRR, infatti, il Ministero gestisce quella missione, ma entro la fine di febbraio 2026 dovranno attuare quei progetti e rendicontarli con tutte le spese previste. Tenuto conto che l'erogazione di quei finanziamenti avviene per *tranche*

contratti. Questo meccanismo di finanziamento messo in campo dal Governo e le incertezze sulla rimodulazione del PNRR aggravano ulteriormente questa particolare condizione, soprattutto per gli atenei più piccoli e più giovani. Diciamo chiaramente che le misure di questo decreto-legge, nato per fronteggiare le emergenze, costituiscono rattoppi per far fronte soltanto alla punta dell'*iceberg* dei problemi che siamo chiamati a gestire. Sarà un fallimento: lo sarà per il centrodestra, ma, prima ancora, lo sarà per l'intero Paese, signor Ministro. Non ci sarà, dopo il vostro fallimento, un altro PNRR. Ci saranno costi drammatici per l'Italia intera. Il Piano è un'opportunità di quelle che non passano mai due volte nello stesso secolo. Non è casuale che qualcuno si sia spinto a paragonarlo al Piano Marshall, l'unico provvedimento, nell'intera storia italiana che, nel secondo dopoguerra del Novecento, sia riuscito a ridurre il divario sia riuscito a ridurre il divario tra il Nord e il Sud del Paese. Ecco perché, ancora una volta, state perdendo una grande occasione. Solo che, questa volta, la perdita di questa grande occasione la pagheranno le nuove generazioni e l'Italia intera.

oggi, come sapete, l'Aula è chiamata a convertire il decreto-legge che introduce disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza: un piano fondamentale, un piano strategico per il futuro della nostra Nazione.

prevede una sostanziale revisione del sistema di *governance* del PNRR, il rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti chiamati ad attuare gli interventi previsti dal PNRR e dal PNC, l'accelerazione e la semplificazione delle procedure PNRR in vari settori e l'attuazione delle politiche di coesione, di politica agricola comune e di politica giovanile. L'intento, come abbiamo ribadito più volte, è quello di snellire le procedure per accelerare gli investimenti e i cantieri, dando piena attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza, con una particolare attenzione alle materie di fondamentale importanza per lo sviluppo nazionale, quali l'ambiente, l'energia, l'edilizia scolastica e le infrastrutture. Desidero sottolineare l'apprezzabile lavoro che è stato svolto dalla Commissione bilancio, da tutti i colleghi,

con grande orgoglio che, anche grazie a un clima collaborativo, partecipativo e - come ha detto prima il collega Gelmetti - anche ordinato, è stato possibile migliorare in alcune sue parti il testo originario, grazie anche alla collaborazione di tutti i membri del Governo, che sono sempre stati presenti ai nostri lavori di Commissione. Noi oggi raccogliamo il frutto di quella che è stata una vera e propria maratona di audizioni, con un lavoro sinergico tra amministrazioni competenti, portatori di interesse e rappresentanti degli enti locali e delle Regioni, in una continua interlocuzione con i rappresentanti del Governo, ma anche con un approccio non ideologico al PNRR da parte dei Gruppi di maggioranza. Molto lontano, invece, da ciò che avveniva in passato e altrettanto estraneo alle continue proprietà intellettuali e politiche rivendicate sul tema da alcuni Gruppi presenti in quest'Aula. A noi interessa altro. A noi interessa condurre in porto il PNRR, evitando gli sprechi e garantendo la realizzazione di opere utili, che abbiano cioè la legittima prospettiva di produrre crescita e ricchezza, volano dell'Italia del futuro.

C'è stato l'intervento per le imprese esecutrici e i subappaltatori, già gravati dal caro delle materie prime, che potranno accedere alle anticipazioni del sistema creditizio in tempi più rapidi, evitando criticità di cassa. La modifica infatti consentirà loro di emettere la fattura relativa ai lavori riportati in SAL anche in assenza del relativo certificato di pagamento; un'agevolazione che indubbiamente contribuirà a dare più solidità al sistema. poi il ruolo centrale delle comunità energetiche rinnovabili (CER), riconosciuto alle imprese artigiane, e le semplificazioni relative agli impianti a energia rinnovabile. Ricordo in questo senso, nel rispetto di determinate soglie in aree classificate idonee, l'esclusione dalla valutazione di impatto ambientale del fotovoltaico, degli impianti di stoccaggio da fonti rinnovabili, del ripotenziamento di impianti eolici esistenti e dei piccoli impianti marini dal piano di gestione dello spazio marittimo. il potenziamento e l'affinamento delle attività di controllo degli incentivi Transizione 4.0. Ci sono gli interventi di velocizzazione dei pagamenti della pubblica amministrazione, con l'efficientamento dei processi di spesa e l'introduzione di obiettivi annuali di rispetto dei tempi di pagamento per i dirigenti responsabili. poi la nomina di un commissario straordinario, a cui ha accennato prima la relatrice Testor, anche per garantire la realizzazione della linea 2 della metropolitana di Torino.

con profondo rammarico che questo tema è quotidianamente oggetto della più bieca strumentalizzazione politica e lo è stato anche poco fa in quest'Aula. In particolare faccio fatica a digerire la narrazione, da parte di alcuni Gruppi, secondo cui il Governo starebbe improvvisando e non sarebbe in grado di mettere a terra le infinite potenzialità del Piano di ripresa e resilienza. Per rispondere a chi accusa il Governo Meloni di disperdere e sprecare il grande risultato europeo ottenuto dal presidente Conte, voglio ricordare che il PNRR fu tutt'altro che un successo negoziale, ma la mera certificazione dell'Italia come fanalino di coda dell'Europa in fatto di crescita e occupazione. *(Applausi)*. Fu su questi parametri che i fondi vennero allocati. Se proprio ci tenete tanto, onorevoli colleghi, ve lo concediamo: grazie per aver ammorbato l'economia italiana nell'ultimo decennio! *(Applausi)*. A chi fa della gratuità il proprio *mantra* - era gratis il superbonus, era gratis il reddito di cittadinanza, ora è gratis il PNRR - ricordo che che più di 120 miliardi di euro del PNRR sono a debito, che solo sette Paesi europei hanno richiesto la propria quota di prestito e che solo tre - Romania Grecia e, appunto, Italia - hanno applicato la formula del tutto e subito. Magari, al netto dei pruriti da convenienza elettorale, un approccio maggiormente prudenziale sarebbe stato più opportuno, soprattutto in assenza di piani credibili per mettere a terra le opere in tempi utili.

sugli eventuali effetti economici moltiplicatori riferibili ad opere come camposanti e loculi, progetti di *bike sharing* in contesti bucolici, riparazioni parafulmini, bocciodromi o case di nuova socialità e accoglienza di di popoli in transito. Stiamo scrivendo le pagine dell'Italia del domani e il termine Next generation EU, onorevoli colleghi, dovrebbe suggerirci qualcosa al riguardo. Oppure qualcuno preferisce non sporcare la favola del Governo dei migliori? Allora continuiamo a scrivere un'altra pagina, che è quella dell'Italia di oggi. concludendo, come già accaduto su altre partite, il Governo Meloni e le forze politiche che lo compongono sono al lavoro, con grande senso di responsabilità e consapevolezza istituzionale, per mettere ordine, per semplificare, per velocizzare i processi, creando le condizioni per la piena realizzazione del PNRR. Sarà un percorso lungo e sono sicura anche molto complesso, ma che grazie alle riforme oggi introdotte potrà registrare dei miglioramenti significativi. Quello che chiediamo è di votare convintamente il provvedimento in esame e, a chi ha contribuito a creare queste criticità, non solo chiediamo di non emettere dei giudizi sterili e infondati, ma soprattutto di non fomentare allarmismo e catastrofismo per un bieco tornaconto elettorale.

del Governo, oggi fingerò di essere ancora sindaco del mio Comune e di essere per una qualche ragione audita nell'Aula del Senato; farò quindi un intervento da sindaco raccontandovi come percepisco il vostro decreto-legge sul PNRR. Parto dalla seguente riflessione. Quando nei corridoi del Senato mi confronto con altri senatori che sono o sono stati sindaci percepisco che, come me, valutano l'efficacia dei provvedimenti pensando all'organizzazione dei Comuni, alle competenze dei sindaci, alla capacità amministrativa.

nazionale dei Comuni d'Italia intorno ai 40 miliardi, un quinto dell'intero piano), eppure non si parla di capacità amministrativa dei Comuni. Il decreto-legge si occupa di sopprimere le agenzie governative e di riorganizzare funzioni statali. Come è possibile, perché? Vi racconto cosa succede nei Comuni. Ci sono Comuni del centro della Sardegna in cui un geometra (molto più raramente un ingegnere) molto spesso vicino alla pensione è a capo degli uffici tecnici di tre Comuni; ci sono Comuni in cui il geometra di cui sopra è l'ufficio tecnico; ci sono Comuni con tre dipendenti; abbiamo segretari comunali piemontesi che gestiscono una decina di Comuni in montagna. Tantissimi sono i Comuni che vedono i propri uffici svuotati da procedure di mobilità e concorsi in favore delle Regioni che pagano meglio (in effetti i dipendenti comunali sono anche sottopagati) e che li espongono a minori

dovremmo parlarne a proposito del PNRR, che - lo ripeto - per un quinto è in capo ai Comuni. Del resto tutti noi ricordiamo le parole profetiche di Draghi ai sindaci: il successo del PNRR è nelle vostre mani. Già allora, senza strumenti e regole chiare, suonava un po' minaccioso, oggi sembra una bella presa in giro. Voi invece parlate di *governance* centrale, di Agenzia per la coesione territoriale, di Dipartimento per le politiche di coesione. Vi do una notizia: nessun responsabile di procedimento di un Comune si preoccupa di sapere se chi risponde da Roma ai quesiti sul PNRR sia l'Agenzia di coesione territoriale o il Dipartimento per le politiche di coesione. Si preoccupa soltanto dalla risposta efficace e del supporto vero che vorrebbe ricevere. grottesco. Parafrasando la regina Maria Antonietta, presidente del Consiglio Meloni, i Comuni hanno bisogno di aiuto, sopprimete l'Agenzia di coesione territoriale.

Di fronte a questi ritardi il vostro asso nella manica è modificare la struttura di *governance* di Palazzo Chigi, anziché operare una vera, effettiva, urgente, improrogabile Non si capisce poi in quale modo la nuova struttura dovrebbe essere maggiormente funzionale agli obiettivi prefissati e superare così gli ostacoli che voi stessi lamentate. Non lo capiamo noi del MoVimento 5 Stelle (poco male), ma sembrano non capirlo nemmeno gli stessi tecnici e questo preoccupa preoccupa decisamente un po' di più. Altro tema è il tempismo con cui mettete mano alla *governance* delle politiche di coesione. Sono tre le grandi perplessità davanti a questa tempistica. luogo, questo è l'anno cruciale del PNRR, quello in cui la maggior parte degli interventi deve essere messo a terra; in secondo luogo, è l'anno in cui il ciclo di programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali entra nel vivo; è l'anno in cui - si spera - dovranno essere ripartite le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027. Dico che si spera perché ancora nulla si muove su questo fronte. Mesi fa ho anche presentato un'interrogazione al ministro Fitto, ma ancora attendo risposta. Il metodo utilizzato per affrontare l'urgenza sembra essere quello di creare un'altra emergenza. Eravate pronti: sì, insistiamo, perché con questo *slogan* avete trasmesso tanta fiducia. Ma pronti a cosa? Non c'è un tema, dico uno, che state affrontando con la disinvoltura di chi è pronto. I sindaci, da chi si è dichiarato pronto, si aspettavano sicuramente altro, ad esempio la previsione di un'assistenza tecnica con esperti qualificati che vada effettivamente a supporto dei Comuni, che sono attuatori di interventi del PNRR, anche quelli più periferici, per la scelta delle procedure, la predisposizione degli avvisi, la gestione degli interventi, il monitoraggio e il controllo. Si aspettavano il potenziamento del Fondo progettazione, l'incremento delle risorse e ancora più semplificazioni nelle procedure. Sarebbe stata gradita la possibilità per i Comuni di bandire le progettazioni prima di avere disponibili le risorse per le opere, perché soltanto così sono in grado di avere quelle benedette opere immediatamente cantierabili, che sono suscettibili di finanziamento nella maggior parte degli avvisi PNRR e delle politiche di coesione. riguarda i sindaci. Da senatrice, invece, dovrei dirvi altre cose. Vorrei ad esempio ricordare che semplificazione e deregolazione non sono sinonimi, e scegliere di non sottoporre a valutazione di impatto ambientale qualsiasi impianto fotovoltaico con una potenza fino a 30 potenza fino a 30 kilowatt che sia sito in un'area idonea non è semplificare: è pericoloso. Dovrei ricordarvi che la VIA serve proprio per garantire che tali impianti non abbiano degli impatti pregiudizievoli di interessi pubblici fondamentali, come la tutela del patrimonio ambientale, di quello paesaggistico e il rispetto delle comunità Concludo, signor Presidente. Il Next generation EU, da cui il nostro PNRR discende, è nato da una visione europeista forte, come poche volte si era visto dalla nascita delle istituzioni comunitarie. È nato grazie ad uno sforzo di unità in cui l'Italia, con il presidente Giuseppe Conte, ha saputo per la prima volta da tanto tempo *leadership* e credibilità internazionale. Il PNRR e le politiche di coesione hanno nella coesione il principio più forte: la riduzione del divario tra Nord e Sud dell'Europa e del nostro Paese (articolo 119 della Costituzione). Se una sola cosa, tra le tante sbagliate, potessimo vedere modificata nel vostro decreto-legge, quella è l'eliminazione della totale ambiguità sulla destinazione delle risorse non spese del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020.

Grazie, Presidente. membri del Governo, onorevoli colleghi e colleghe, c'è un po' di amarezza nel trattare questa tematica, non tanto sul merito del provvedimento o sul tema generale del PNRR, ma per l'atteggiamento delle opposizioni.

cosa accada. Ma questo tipo di atteggiamento il Governo non l'ha avuto. Anzi, ha detto: siamo pronti a collaborare e lavoriamo per cercare di risolvere i problemi. Questo è stato l'approccio. Invece, dall'opposizione

principali oggetto di scontro e di battaglia politica. Ma il Piano di ripresa e resilienza, che riguarda tutti e dovrebbe darci la prospettiva del futuro sviluppo del Paese, dovrebbe però quanto meno portarci ad una discussione più seria. Il ministro Fitto avrebbe potuto dire che, di solito, quando si fa un piano, si parte dai progetti di sviluppo che si hanno e poi si chiedono i soldi;

la quantità della spesa che dà l'idea di un'economia che si può riprendere a lungo termine, ma, casomai, è la qualità degli investimenti che possono generare prodotto interno lordo, da cui si può misurare effettivamente lo sviluppo a lungo termine di un Paese.

ma probabilmente a causa di una politica di *austerity* che l'Europa porta avanti da più di vent'anni, sulla quale noi ci siamo sempre battuti.

a maggior ragione nei Comuni del Sud, cui è destinata una buona parte del Piano. Queste cose però il Ministro e il Governo non le hanno dette; potevo dirle io politicamente, ma non le abbiamo dette. Il Ministro ha detto che noi siamo pronti a fare che cosa? Sappiamo da sempre che l'Italia

improvvisamente tutti diventiamo efficienti da un giorno all'altro. No, questo è il risultato vero che dobbiamo mettere in evidenza. Sapevamo già che c'era questa parte di soldi che probabilmente avremmo fatto fatica a spendere. Qual è allora il ragionamento del Governo? Quello

modo di pensare che sicuramente andranno a buon fine e genereranno prodotto interno lordo che ci servirà per poter poi pagare gli interessi della maggior parte dei prestiti. Vorrei infatti sottolineare che due terzi di queste risorse infatti non sono regalati,

Si metteva in discussione l'Europa solo alzando la manina per dire qualcosa. Oggi, finalmente, si prende coscienza che non erano proprio tutti soldi regalati; bene, un passo in avanti l'abbiamo fatto. questa è la strada che il Governo deve giustamente mettere in campo. Ragioniamo insieme allora su quali sono le opere su cui poter girare i soldi, sapendo che ragionevolmente potranno essere portate Per esempio, una parte della minoranza - è arrivata da Calenda questa proposta - ha detto che si potrebbero spostare delle risorse sugli

che dovrebbe animare tutti noi in maniera costruttiva e seria. Invece, come sempre, c'è la solita questione: «Brutti, cattivi, non volete prendere i soldi; adesso ci portate al fallimento. Siamo stati bravi noi». Posso dire che effettivamente in questa Nazione un po' di infantilismo politico

che non ci possiamo permettere è pagare gli interessi su mutui accesi per opere che non realizzeremo mai? Su questo siamo d'accordo tutti quanti? *(Applausi)*. Sarebbe una follia.

Poi il Governo farà di tutto per spendere i soldi, cercando ovviamente di orientarli, verificando alcune gare andate deserte. Insomma, se fai una gara sui treni a idrogeno e vedi che non partecipa nessuno, magari può essere che non sia proprio lo strumento ideale per creare sviluppo in questo Paese; magari orientiamoci su qualcosa di differente. Questo è il nostro intervento dal punto di vista politico, con la speranza davvero che si possa ragionare in termini seri. Mi avvio

cosicché a comandare l'Italia saranno le istituzioni europee e non invece un Governo legittimamente votato dagli italiani. Grazie, Presidente. stiamo affrontando il tema del PNRR all'insegna di una grande responsabilità. Sappiamo che è un piano che non abbiamo scritto noi e che forse, non solo non abbiamo ideato, ma per alcuni aspetti in verità non avremmo assolutamente ideato così; anzi, riteniamo che per molti aspetti non ci siano elementi di corrispondenza a quelle che sono priorità

proprio con l'obiettivo di mettervi mano, di renderlo il più possibile cogente e, soprattutto, di non perdere assolutamente neanche un euro delle risorse e dei finanziamenti

sul quale sono molto lieta che si stia ponendo grande attenzione, anche nei rapporti con l'Unione europea. Crediamo infatti che sia assolutamente fondamentale preservare l'ambiente e la natura,

sulle case *green*, che sinceramente riteniamo che poco si addica al nostro tessuto di piccole proprietà a livello nazionale. Ci sono anche elementi di riforma molto rilevanti sui quali si deve operare: penso alla riforma della pubblica amministrazione - sono stata per anni un assessore, prima, un consigliere di Roma Capitale poi - di istituzioni, di enti locali, e ben sappiamo quanto è

Non è una sfida semplice quella che il Governo ha voluto attribuire al nostro qui presente Ministro. È una sfida da far tremare le vene nei polsi, e devo dire che questo strumento

e poi, in un secondo momento, quando avremo rivisto la *governance* e avremo semplificato e snellito ulteriormente le procedure complesse e farraginose, potremo, forse, cominciare a fare un'analisi sui tempi e sulle eventuali critiche. Vediamo insieme le parole d'ordine che sono state redatte in questo decreto-legge che ci apprestiamo a convertire: snellimento delle procedure; semplificazione e presa d'atto delle difficoltà di una macchina amministrativa, come dicevo, assolutamente complessa; flessibilità, che è stata oggetto di azioni abbastanza serie e perentorie da parte del Ministro e del Governo nei rapporti con l'Unione europea, una flessibilità urgente; l'adozione di una politica dei vasi comunicanti, per cui se un fondo può essere utile per altro, magari perché, come diceva chi mi precedeva, un'opera non è realizzabile, ebbene, che si possa comunque utilizzare nel miglior modo possibile, con una messa a terra adeguata.

bilancio del Senato, nella quale mi onoro di poter operare, sia nel lavoro svolto dal Governo nel redigere il decreto-legge medesimo. Mi riferisco allo spirito di squadra. Quando parlo di squadra intendo squadra Italia: ognuno di noi veste i panni di un esponente italiano. Oltre a questo, vorrei richiamare anche un altro spirito: quello del senso di responsabilità che ciascuno deve avere.

Perché lo spirito è quello di subentrare là dove c'è una difficoltà, in ambito amministrativo, nella realizzazione di uno di questi piani o di una di queste missioni. Quindi, il Consiglio dei ministri per primo si assumerà questa responsabilità, ma quest'ultima poi ricadrà ovviamente su quei Comuni, su quegli enti locali, su quegli assessori e su quei dirigenti che dovranno andare a realizzare tutto ciò che noi oggi voteremo in questa Aula. Per questo li dobbiamo sostenere. sostenere. Rivendico con favore, per esempio, il fatto che si scelga di assumere più personale nella pubblica amministrazione *(Applausi)*, perché abbiamo bisogno di una pubblica amministrazione efficiente, ma con blocchi del *turnover* di anni è difficile che possano essere efficienti.

diventare più produttivi con le risorse messe a nostra disposizione, in termini di opere pubbliche realizzate, grazie a politiche di incentivi, nelle quali noi crediamo fermamente.

orgogliosi quando - prima qualcuno richiamava la sanità - avremo stipendi più alti per i medici; saremo tutti orgogliosi se riusciremo a mettere bene a terra questo PNRR. Ognuno deve vestire il vestito del membro della squadra, dal più piccolo consigliere comunale al più alto dirigente della nostra Nazione, perché abbiamo veramente l'opportunità, grazie a questo Piano, di far crescere ulteriormente la nostra Italia. Signor Presidente, parlerò dei ritardi nell'implementazione del PNRR. Quando si parla di ritardi spesso ci si riferisce ai ritardi nella spesa, però dobbiamo ricordarci che il PNRR è fatto di due componenti: le riforme e la spesa. Attenzione: le riforme sono almeno tanto importanti quanto quanto la spesa. È stato calcolato che metà dell'impatto sulla crescita della produttività del PNRR viene dalle riforme e il resto viene dalla spesa.

l'introduzione dei decreti che sono necessari per l'attuazione della riforma Cartabia, che ora sono rinviati a fine anno. Ricordiamoci che qui c'è un obiettivo molto preciso: entro la fine del 2026 dobbiamo ridurre i tempi della giustizia civile del 40 per cento, il che ci porterebbe un po' più vicini alla media europea ed è fondamentale. Sappiamo che il ministro Nordio presenterà nuovi atti di riforma e siamo in attesa, però c'è una questione di urgenza in quest'area. C'è una questione di urgenza anche nella seconda area di cui volevo parlare, quella della concorrenza. alla legge annuale sulla concorrenza, sappiamo che il Governo vi sta lavorando. Secondo la stampa doveva essere presentata in qualche Consiglio dei ministri passati, ma non è ancora avvenuto. Devo essere sincero su questo: ho l'impressione che alcune forze della maggioranza non credano completamente nell'importanza della concorrenza per l'economia italiana. Forse mi sbaglierò, però assistere a certe discussioni sui balneari, sui taxi e così via mi ha fatto venire il sospetto che ci sia un po' di

che davvero non riesco a spiegare, perché ritarderanno - per lo meno in termini di implementazione - il PNRR. Mi riferisco, in particolare, alla decisione di cancellare territoriale e di trasferirne le responsabilità a un Dipartimento della Presidenza del Consiglio. È chiaro che questo nell'immediato crea dei ritardi. C'è poi un'area che - vorrei sottolineare - non è stata trattata abbastanza dai precedenti Governi e mi sembra neanche da questo Governo

ma alla creazione di adeguati incentivi perché chi sta nella pubblica amministrazione si senta motivato a fare il suo dovere. Questo significa fissare degli obiettivi che devono essere raggiunti, monitorarne il raggiungimento e poi premiare chi se lo merita e non premiare chi non se lo merita, invece di dare

L'ultima area di riforma è quella che possiamo definire la madre di tutte le riforme: quella del fisco. Per questo c'è la legge delega, anche se devo dire che molte cose nella legge delega ancora non sono chiare, comunque si è scelta questa strada. che anche come contribuente e come cittadino, di fronte ad una riforma del fisco, la prima cosa che vorrei sapere è qual è l'obiettivo in termini di riduzione del carico fiscale e quali sono le fonti di finanziamento. Questi dati non sono scritti nella legge delega. Talvolta si dice che la riforma sarà finanziata con il taglio

Se si vuole ridurre il carico fiscale, si deve tagliare la spesa e non c'è nessuna indicazione di quale spesa sarà tagliata. in volta si trova un modo per finanziare, ad esempio, i tre miliardi, ma si deve avere una prospettiva di medio termine se si vuole fare in modo che il taglio delle tasse abbia un effetto, ad esempio, sulle decisioni di investimento. Venendo alla questione della spesa e degli investimenti pubblici, ci sono dei ritardi, come ci ha detto la

Chiariamo la questione: è vero che nel 2021 e nel 2022 la spesa è stata inferiore a quello che era stato programmato, ma si trattava di importi minori, abbastanza bassi, tant'è vero che la Corte dei conti ha calcolato che per recuperare i ritardi del 2021 e del 2022 sarebbe sufficiente nei prossimi anni, compreso questo, avere una maggiore spesa di 4-5 miliardi, che non è poco, ma rispetto a quello che comunque si sarebbe dovuto fare (40-45 miliardi) miliardi) non si tratta di un aggravio particolarmente forte. Ricordiamo che quegli obiettivi di spesa erano stati fissati con l'approvazione della maggioranza che c'era al tempo di Draghi, che comprendeva anche una buona parte delle attuali forze di maggioranza, perché non è che questi numeri siano usciti soltanto dalla testa di Mario Draghi: sono stati approvati da una

questi finanziamenti sono di importi mai raggiunti da nessun Paese. Anche qui ricordiamo che si tratta di tornare a un rapporto tra investimenti pubblici e PIL che c'era in Italia vent'anni fa. Quindi, non è una cosa che non è mai stata fatta. Si dice che non c'è più personale compreso nei Comuni. Anche qui, chiariamo i numeri. Tra il 2008 e il 2020 il personale della pubblica amministrazione si è ridotto del 7,7 per cento, non del 30 per cento. Ricordiamo che in questo periodo molti Comuni hanno aggirato i vincoli al personale creando una marea di società partecipate. Quindi, l'occupazione della pubblica amministrazione non è scesa così tanto come alcuni sostengono. Si dice che anche questo è debito. Non venite a dirlo a me, che sono sempre preoccupato del debito pubblico, ma ricordiamo una cosa: il debito pubblico è creato dal *deficit* pubblico ed il *deficit* pubblico è fissato anche in base a motivi macroeconomici. Il DEF di ieri ha fissato un obiettivo, un sentiero per il *deficit* pubblico e quindi per l'accumulazione di debito. Il che vuol dire che, se spendiamo meno i soldi del PNRR, dato quell'obiettivo di *deficit* macroeconomico, dobbiamo spendere di più in qualcos'altro; e se spendiamo di più in quel qualcos'altro, però a finanziare quel qualcos'altro a un tasso di interesse molto più alto di quello che si paga, invece, sui fondi del PNRR. Si tratta di un prestito agevolato e questo dobbiamo ricordarcelo.

servirà per la transizione. Vi sono altri due mesi per l'implementazione dei decreti per attuare la riforma. Si arriverà a metà giugno e avremo passato diversi mesi,

sui possibili cambiamenti che il Governo vuole effettuare. Non sappiamo bene quali siano questi cambiamenti, ma è chiaro che, finché si discute, anche qui non si sta progredendo in quello che dovremmo fare. In conclusione,

credo che oggi sia fondamentale riconoscere la grandezza del lavoro svolto, sia dal Governo che dalle Commissioni per quanto di loro competenza, perché questo disegno di legge segna veramente un passo fondamentale. Sì, l'orizzonte del 2026 non è lontano. Lo sappiamo e abbiamo il dovere di agire, affinché quello che oggi sembra un limite temporale a dir poco minaccioso diventi un termine naturale entro il quale mettere a terra le risorse del PNRR, per trasformarle in progetti concreti e non bocciodromi o partite e tornei di briscola. *(Applausi)*. *Governance,* burocrazia, situazione degli enti locali, in particolar modo in materia di personale qualificato, aumento verticale dei costi e risorse effettivamente spese rispetto a quelle preventivate. Queste, signor Presidente, sono le principali criticità, purtroppo profondamente connesse tra loro, che il Governo si è trovato ad affrontare. Ma con responsabilità, concretezza e coerenza (e sottolineo l'elemento della coerenza), questo Governo ha operato una completa rivisitazione del sistema dei procedimenti, partendo da uno stato di fatto che nulla aveva a che fare con quanto tanto decantato dal precedente Governo. Siamo entrati in corsa; c'è ancora molto da fare e molto terreno da recuperare. Ma questa è una sfida che siamo determinati a vincere. Vorrei fare un esempio: si pensi a una scala, con dei valori che vanno da 0 a 100. Noi pensavamo di entrare al punto 6? No, cari colleghi, siamo entrati al punto 2. Presidente,

Abbiamo affrontato la criticità della *governance*, una bella parola, che pochi prima di noi avevano capito fino in fondo. È fin troppo chiaro quanto sia stato e sia importante lavorare sul principio della semplificazione, ma anche della certezza. Questo Governo e questa maggioranza hanno agito perché tutto quello che nei piani precedenti doveva essere semplificazione si era invece trasformato in una vera e propria trappola: tonnellate di carte e grande burocrazia avevano messo a repentaglio il raggiungimento dei traguardi. Signor Presidente, sempre ai colleghi dell'opposizione vorrei ricordare che questa criticità non è emersa oggi o negli ultimi sei mesi, ma è emersa

di un piano a scatola chiusa, di un piano basato sì su principi condivisibili, ma per i quali sarebbe stato impossibile dare un giudizio. Ricordo nuovamente le sue parole: se non so come si intendono perseguire quegli obiettivi, come facciamo ad approvarli? Oggi, con questo decreto a supporto della *governance*, riusciamo a fare grandi interventi; lo dico come tecnico e voglio citarne alcuni, già

della struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio, un organo fondamentale per il monitoraggio (finalmente si parla di monitoraggio) e l'attuazione del piano stesso, a garanzia del corretto svolgimento di tutte le istruttorie relative alle proposte di aggiornamento. La stretta sul rispetto dei cronoprogrammi prevede l'eventuale nomina di amministratori terzi o commissari in caso di inerzia o di difficoltà tecnica degli enti attuatori, per portare avanti le progettualità esecutive. Noi vogliamo portare i progetti fino in fondo e non lasciarli a metà, come è stato fatto fino ad oggi. Le disposizioni di controllo e monitoraggio degli interventi finanziati permettono di verificare l'efficacia e la legittimità dei vari *step* programmatici. C'è poi la famosa semplificazione delle procedure di gestione finanziaria, attraverso lo snellimento dei criteri di versamento sui conti correnti, che fino ad oggi avevano bloccato intere aziende. Oltre a tutto questo, al Governo va dato il merito di aver fatto anche il codice degli appalti, snellendo le procedure.

è quella in cui versano gli enti locali per quanto riguarda il personale qualificato. Parlo di tutti quei Comuni soggetti attuatori che sono privi delle professionalità, delle conoscenze e delle abilità necessarie a mettere in pratica i vari progetti secondo i dettami del PNRR. La maggior parte ha dovuto fare i conti microdisposizioni, circolari, a volte in contrasto tra di loro; addirittura dei progetti hanno ricevuto pareri negativi o contrastanti tra loro in corso d'opera, quando già era quasi pronta la parte dell'autorizzazione definitiva. Io ho parlato con i miei tecnici, i quali mi hanno detto che reclutare personale a tempo determinato ha grossi limiti a livello pratico. Una persona, seppur qualificata, una volta assunta deve prima capire come funziona la macchina amministrativa, poi deve realizzare il progetto, lo deve contestualizzare rispetto alla realtà e ai luoghi e infine deve tener conto dei dettami del PNRR. Ricordiamoci che i dettami non sono gli stessi; in questi mesi sono cambiati a causa delle disposizioni, delle micro-disposizioni e di varie circolari che ne hanno via via via mutato il modo di essere non solo applicati, ma purtroppo anche interpretati. Finisce il tempo e i Comuni che fanno? Si trovano sprovvisti di personale, perché è finito il tempo. Quella persona qualificata

il problema e dando un ulteriore segnale di concretezza e di reale supporto ai Comuni, oltre a contrastare il fenomeno del precariato. Basta *slogan*: noi lo facciamo! Quindi, chiedo a chi oggi strumentalmente attacca il Governo come sia possibile pensare che, senza la revisione critica fatta dal disegno di legge in esame, si potesse arrivare a dama entro i limiti stabiliti. L'ultima cosa che voglio evidenziare è l'aumento dei costi, sia delle materie prime sia delle parcelle dei professionisti. Viviamo in un mondo completamente diverso rispetto a quello del 2021 e chi non se ne è reso conto forse vive sulla luna oppure non ha mai pagato una bolletta o non ha mai raffrontato la bolletta di due anni fa con quella di oggi. Ecco perché dico che il Governo, con l'articolo 7, è intervenuto efficacemente, togliendo questa criticità. Signor Presidente, concludendo, era necessario prendere atto di queste difficoltà oggettive e il Governo di centrodestra l'ha fatto. Pensate che in due mesi ha portato avanti 30 traguardi necessari per richiedere la terza rata. Il Governo Draghi ne aveva realizzati 25 su 55, in dieci mesi. In due mesi,

a cui poi rispondono il ministro Giorgetti, che vuole spendere tutti i fondi del PNRR ma con un po' di flessibilità, o il ministro Fitto, che vuole spostare i fondi dal PNRR ai fondi strutturali per avere maggiore flessibilità e più tempo.

eliminare il divario esistente tra le zone interne e il resto del Paese e tra i cittadini, per non creare cittadini di serie A e di serie B. Qui servono gli asili nido, serve rinforzare il personale della pubblica amministrazione e servono investimenti

tra poco ci accingeremo a votare la conversione in legge del decreto-legge recante disposizioni urgenti volte a favorire l'attuazione del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari, nonché misure per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Le numerose audizioni che si sono tenute in Commissione - rispetto alle quali colgo l'occasione per ringraziare gli auditi per il prezioso contributo che hanno fornito hanno fotografato le aspettative relative al PNRR accomunate dalla richiesta di semplificazione, efficienza e rapidità necessarie per dare attuazione a tutti quei progetti che potranno assicurare all'Italia Le risorse messe a disposizione del nostro Paese rappresentano certamente una possibilità per il futuro dell'Italia, ma anche una grossa responsabilità nei confronti delle future generazioni. Il loro investimento deve essere mirato e oculato, in quanto una parte delle risorse è sì a fondo perduto, ma una parte altrettanto significativa rappresenta invece un debito da restituire e, quindi, per essere ripagato, deve avere un congruo ritorno economico. due anni di distanza dalla presentazione del piano è a tutti evidente la necessità di un'azione di forte semplificazione e di snellimento delle procedure, al fine di non compromettere l'efficienza degli investimenti. Le difficoltà nell'attuazione degli interventi sono certamente dovute a diversi fattori, quali i rincari delle materie prime e dei prodotti energetici emersi a partire dalla fine del 2020 e acuiti con lo scoppio della guerra in Ucraina. Essi hanno determinato uno slittamento in avanti dei cronoprogrammi e degli investimenti, a cui vanno aggiunte le difficoltà delle amministrazioni pubbliche, fortemente depotenziate dopo anni di blocco del *turnover,* che lamentano seri problemi di personale. In modo particolare lo riscontriamo nei piccoli Comuni, che faticano a predisporre le progettazioni degli interventi, le gare e a seguire i lavori a causa della difficoltà di reperire tecnici esterni, anche a seguito del mercato drogato dal superbonus. Né i Comuni hanno disponibilità di loro tecnici in organico. In ultimo - ma non per importanza - i tempi di realizzazione impiegati nel nostro Paese per un'opera pubblica appaiono incompatibili con la scadenza del 2026 del PNRR. È doveroso ricordare che in Italia occorrono mediamente più di quattro anni per realizzare un'opera pubblica e che per quelle al di sopra dei 100.000 euro arriviamo addirittura a sedici anni. L'impostazione generale del decreto-legge va proprio nella direzione di semplificare e migliorare i processi di attuazione e *governance* del PNRR, nonché le politiche di coesione, di accelerare e snellire le procedure, specie con riferimento all'affidamento dei contratti pubblici PNRR e al PNC. Nello specifico prevede la revisione della *governance,* il rafforzamento della capacità amministrativa e lo snellimento delle procedure, il potenziamento delle politiche di coesione anche in un'ottica di integrazione con il PNRR.

detto dal collega Lombardo, si tratta non di piegarsi alle piccole richieste delle corporazioni, ma di avere il quadro certo e di sapere se la risorsa naturale della spiaggia è o meno scarsa e quindi se la direttiva Bolkestein è applicabile o meno. Allo stato attuale,

tutto e il contrario di tutto, visto che anni addietro non era a favore dell'opera. Collega, meglio cambiare idea su un ponte che mandare a processo un Ministro, con il rischio di quindici anni di galera, e non perché era contrario ai decreti sicurezza di allora - ancora oggi, infatti, troviamo le foto di Conte che li pubblicizza come traguardo raggiunto - ma solo per il fatto di non essere più alleati di Governo: questo è molto grave. Tornando al merito del decreto-legge in discussione, sono felice che sia stato accolto l'ordine del giorno a mia prima firma, che prevede nell'ambito del settore marittimo, portuale e logistico, in coerenza con gli obiettivi relativi alla decarbonizzazione del settore, iniziative governative utili al rinnovo e al *refitting* di navi adibite ad attività crocieristica. L'importanza di poter ricevere nei porti navi da crociera che abbiano il minor impatto ambientale possibile - lo dico da spezzina - può realmente fare la differenza. In questo le istituzioni possono dare il loro contributo sostenendo gli sforzi del settore nell'uso di carburanti alternativi, sicuri e utilizzabili su larga scala, nonché sostenendo il processo di transizione di tutte le navi, semplificando ed ampliando il Fondo complementare al PNRR per il rinnovo e il *refitting* della flotta mercantile, allargandolo anche a quello delle navi da crociera. una risposta anche a questo settore e, quindi, al turismo nonché all'ambiente, in un'ottica di prosperità e sostenibilità. *(Applausi)*.

alla tempestività di questo decreto-legge e alla necessità di mettere mano, per quanto possibile, a ogni correzione che snellimento delle procedure e sia capace di far rispettare i tempi previsti da una *governance* del PNRR che non ci appartiene e che ci è stata lasciata in eredità - quella sì dai precedenti Governi. La tempestività con cui questo Governo si è immediatamente impegnato nel dare corso agli adempimenti per l'attuazione del PNRR è testimoniata da un bilancio

e il Governo Meloni in soli due mesi conseguire i restanti trenta. I numeri non sono interpretabili. Anche per chi è discalculico è facile capire quello che ha fatto il Governo Meloni rispetto alla alla convinzione di non perdere neanche un solo euro rispetto alle misure e ai finanziamenti previsti nell'ambito del PNRR. Quindi, massimo plauso rispetto a quello che si sta facendo. Un esempio per tutti è la possibilità della stabilizzazione del personale precario, prevista dalle procedure di attuazione del PNRR e che viene anticipata

Quindi tutto quello che l'Italia poteva fare, per mettersi nelle condizioni migliori per adempiere alle scadenze e alle misure previste - ripeto - da un cronoprogramma che non ci appartiene, l'ha fatto.

del Senato della Repubblica ha deciso di avviare un'indagine sulla capacità di spesa e di trarre le risorse disponibili per l'edilizia sanitaria. la necessità ci è stata suggerita da un rilievo della Corte dei conti che mette in evidenza come l'apparato burocratico amministrativo della nostra sanità in oltre trenta anni ha speso, rispetto a 34 miliardi di euro impegnati, non più del 25

il nostro apparato burocratico amministrativo della sanità è riuscito a impegnare 10 miliardi e spenderne neanche il 25 per cento. Ministro, *mutatis mutandis* come dicono quelli più bravi di noi, poveri parlamentari di campagna, che però riusciamo facilmente a fare le dovute proporzioni - se all'articolo 20, in trenta anni, siamo riusciti a raggiungere così importanti

possano essere meglio ritagliate rispetto alle caratteristiche del nostro Paese? Ricordo che non tutti i Paesi dell'Unione europea hanno le stesse caratteristiche e capacità di trarre le risorse, come purtroppo è dimostrato da una lunga

non siamo certo stati noi. Se qualcuno ha tagliato le risorse della sanità dal 2010 al 2019 per 34 miliardi di euro, non siamo certo stati noi. *(Applausi)*. Non è stato certo il Governo Meloni a falcidiare la possibilità di progettazione e di messa a terra dei progetti da parte delle Regioni. Tutti i soggetti che noi abbiamo ascoltato in Commissione, Ministro, sono venuti a denunciare che, ad eccezione di due o tre Regioni, quelle meglio strutturate lascio a tutti i colleghi immaginare quali - la stragrande maggioranza delle Regioni non ha neanche materialmente la possibilità di accedere alle risorse dell'articolo 20,

le risorse già impegnate negli accordi di programma sottoscritti e sottoscrivere nuovi accordi di programma al fine di poter attingere alle risorse che stanno lì, pronte e disponibili, ripeto - ammontano ad oltre 34 miliardi di euro.

dire a chi non riesce ad intendere che noi, almeno sulle tempistiche, abbiamo bisogno di scrivere qualche pagina differente. Voglio sperare ed, anzi, sono assolutamente convinto che lei, che che è riuscito a fare un lavoro così importante, in ambito comunitario riesca a far capire che l'Italia ha tutta l'intenzione di attingere fino in fondo alle risorse, ma che ha bisogno di tempi diversi rispetto alla sua storia, alle sue caratteristiche e a quello che ci consegnano i Governi che ci hanno preceduto fino ad oggi, che hanno letteralmente falcidiato e reso impossibile la capacità delle Regioni di fare progetti e di metterli a terra. *(Applausi)*.

ha dimostrato e squadernato a tutti noi forti disuguaglianze; anzi, ha aumentato quelle già presenti nella società. Da qui si pone dunque la necessità di favorire la coesione sociale perché, se non c'è coesione sociale, è difficile pensare pensare di costruire un Paese che va avanti con una certa forza e determinazione. Questo è il dato e non a caso il PNRR prevede maggiori risorse nel Mezzogiorno.

c'entra poco questo ragionamento. Il tema è se il Paese fa un passo in avanti oppure ne fa uno indietro. Non è nell'ambito della minoranza, dell'opposizione che si sente dire che è quasi un fastidio aver avuto queste risorse.

intervenire, ad esempio, sulla questione ambientale, sulla rigenerazione urbana, sul favorire e costruire anche l'autonomia dal punto di vista energetico; se si opera

di poterli utilizzare. Ma se il messaggio che diamo è che quello che l'Europa ci dice - ad esempio sul terreno *green* - è una baggianata, è chiaro che ci chiederanno conto. Questo è il dato fondamentale; è normale. Io ho

con grande enfasi la maggioranza a cambiare atteggiamento e a smettere di pensare che la colpa è solo di altri. Oggi governate voi vi dovete assumere la responsabilità di fare delle scelte, che però vadano nella direzione di favorire la coesione sociale, che è l'unico modo per per avere davvero una grande forza come Paese. Io sono cittadino del mondo, ma prima di tutto mi sento un brianzolo e non mi vergogno a sentirmi un brianzolo, un italiano e un cittadino del mondo. Il problema è capire se insieme siamo in grado di fare questo e di compiere una

avrò modo di esplicitare in dichiarazione di voto il punto di vista politico sul decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR, nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Riservo questo mio intervento in discussione generale per una riflessione più puntuale sull'incerta capacità di spesa e di messa a terra degli interventi PNRR e PNC da parte dei soggetti attuatori entro il 2026. Esistono difficoltà oggettive e sono note fin dall'approvazione del PNRR nel 2021: tra queste, la capacità di assorbimento degli oltre 191,5 miliardi assegnati all'Italia, quasi un quarto delle intere risorse del Next generation EU. L'Italia è il secondo Paese assegnatario, dopo la Spagna, della parte di risorse a fondo perduto per 69 miliardi, oltre ad essere l'unico ad aver richiesto anche l'intero ammontare delle risorse a debito per 122 miliardi. È stata una scelta ponderata, perché gli investimenti e gli interventi sono stati pensati per dare quella spinta al tasso di crescita del PIL capace di rendere sostenibile il nostro pesante debito pubblico. È stata una precisa scelta macroeconomica. Le ulteriori difficoltà note erano la capacità di assorbimento delle risorse in quelle zone del Paese a bassa dinamica economica e carente specializzazione professionale, nonché la disomogenea efficienza della macchina amministrativa, priva in troppi casi di risorse umane adeguatamente formate per bandi dalla complessità europea e per il rigore della rendicontazione. Il Piano è stato pensato e strutturato anche per essere un'irripetibile *chance* di superare i limiti Paese: spostare in avanti la data in cui affrontarli è stata per anni una rassicurazione, mentre decidere che era arrivato il momento di risolvere è stato un atto di grande maturità collettiva. Non stupisce quindi che i populisti invochino da sempre e tuttora la strategia del rinvio. Deve essere messo in evidenza che, sin dalla campagna elettorale estiva, la propaganda della revisione del PNRR è stato un tema politico sventolato da quelle destre che ancora oggi, a sei mesi dal voto, non hanno saputo esplicitare, come propongono, di revisionare il PNRR. E la richiesta di avere il ministro Fitto in Aula va esattamente in questa direzione, posto che anche l'intervento in occasione della relazione della Corte dei conti sullo stato di attuazione del PNRR non ha chiarito quali siano le intenzioni del Governo. Anche a Bruxelles, dopo aver giustamente chiarito che, una volta rispettati missioni, obiettivi di transizione digitale ed ecologica trasversali e obiettivi trasversali di riassorbimento delle differenze di genere generazionali e territoriali, i singoli progetti possono anche essere sostituiti, sono in attesa di capire cosa propone l'Italia. Il problema della difficoltà di assorbimento delle risorse può essere affrontato in modo serio, e quindi evitando di dire e di agire nella direzione della rinuncia alle risorse per evitare di mettere in crisi la tenuta macroeconomica dell'Italia e invece concentrandosi su due modalità di riallocazione delle risorse. Penso agli interventi massicci per affrontare problemi strutturali come il dissesto idrogeologico, finanziando gli interventi della struttura di missione Italia Sicura, ripristinata proprio con un emendamento dei riformisti al presente decreto PNRR. *(Applausi)* In secondo luogo, penso al rifinanziamento di quegli interventi a capillare capacità di assorbimento come Industria 4.0 *(Applausi)*, capaci al contempo di rispondere ai primari obiettivi di transizione del Piano. del Piano. La messa a terra degli interventi e degli investimenti ritengo necessiti di tre precondizioni: evitare di modificare *governance* e procedure del Piano in corso d'opera; dotare le amministrazioni centrali e periferiche di personale con specifiche competenze e creare strutture di affiancamento per tutti i soggetti attuatori ed in particolare per gli enti territoriali che da soli devono realizzare interventi per 40 miliardi. La riorganizzazione della pubblica amministrazione, il procedere per gli obiettivi - come sottolineato anche dal senatore Cottarelli - e la formazione permanente sono la vera sfida per modernizzare il Paese. La pubblica amministrazione deve tornare ad assumere talenti, deve tornare fra i dipendenti l'orgoglio di appartenenza e il valore di esercitare funzioni pubbliche. Il PNRR è per l'Italia l'ultima, irripetibile occasione di recuperare i *gap* accumulati negli anni. Realizzare il Piano è una priorità che non ha pari. Per questo l'invito al Governo è lasciare da parte le troppe parole e la propaganda e di mettersi al lavoro con grande determinazione. Se questo sarà l'atteggiamento, il Gruppo delle Autonomie non farà certo mancare il proprio fattivo contributo.

il PNRR non appartiene a un Governo: è stato iniziato con il Governo Conte 2, portato a casa fattivamente dal Governo Draghi e gran parte delle opere verrà realizzata da questo Governo e gli effetti per il Paese si vedranno anche nei Governi successivi a questo. l'esigenza e l'importanza di portare a casa i risultati che sono stati proposti con il PNRR sono non di una maggioranza, ma del Paese. Lo dico perché ciò che ha contraddistinto i nostri emendamenti è l'aver portato - da delle soluzioni di semplificazione, ad esempio sulle energie alternative e - dall'altro - di aver dato un contributo, con l'unità di missione Italia Sicura e Industria 4.0, per spendere le risorse del PNRR anche dando una prospettiva

alle aziende che avevano intrapreso un percorso di modernizzazione, ad esempio, di non crollare a causa la pandemia da Covid-19. Dall'altro, con l'unità di missione Italia Sicura, dare risposte ad un Paese fragile da un punto di vista idrogeologico, che però, per una follia della storia, non riesce mai a spendere i soldi per realizzare le infrastrutture necessarie alla sicurezza dei propri territori. La ringraziamo dunque, ministro Fitto, per aver operativamente dato un parere favorevole a questi due emendamenti, che per noi sono un cavallo di battaglia, per averli tolti da un Governo passato, resi attuali e consegnati a una maggioranza che non è

a due emendamenti che mi sono cari e per questo veramente ringrazio il ministro Pichetto Fratin e lei, ministro Fitto. Sì, due Ministri di un Governo che non ho votato, ma che, di fatto, hanno realizzato un piccolo sogno. È dallo scorso Governo che provo a portare a casa un emendamento sul biometano. L'ho redatto insieme all'associazione Elettricità Futura, non mi vergogno di dirlo,

è sempre un modo carino per non dire di no ad una forza che fa parte della maggioranza. Quell'ordine del giorno, però, non ha avuto una conseguenza fattiva. Qui abbiamo invece approvato un emendamento, di Fratelli d'Italia, di Forza Italia e del Terzo polo, che prova a dare giustizia a dare giustizia a chi aveva investito in infrastrutture sul biometano dando corso al PNIEC di Carlo Calenda del 2017. Questi imprenditori si erano poi visti superati, per una diversa interpretazione

un'opera di semplicità. Chi ha rispettato le regole già nel 2017 oggi, finalmente, potrà completare queste infrastrutture. E noi, che abbiamo un disperato bisogno di energia,

che durante la pandemia può aver sofferto più che altre zone del nostro Paese per un blocco improvviso, si sia reso conto delle infrastrutture mancanti. Il PNRR è questo: dare una seconda *chance* al nostro magnifico Paese. Non appartiene a una forza politica, come ho già detto, ma all'Italia. all'Italia. Proprio per questo non ci possiamo permettere di perdere risorse. Se alcuni progetti non sono

materiali e la guerra hanno creato problemi anche ad altri Paesi europei. Sono in molti a chiedere tempi maggiori e un aumento di risorse per quanto riguarda le materie prime. Facciamo squadra in Europa con chi la pensa come noi e con chi chiede più

che questo Paese può fare, anche perché l'Italia ha avuto maggiori risorse rispetto ad altri, proprio perché la pandemia da Covid è stata più difficile. Abbiamo avuto non soltanto più vittime, ma anche una chiusura maggiore rispetto ad altri Paesi. È proprio per questo che l'Europa ci è venuta incontro. Oggi non possiamo far finta di niente e dire che non siamo pronti. Questa è una grande sfida, soprattutto alla pubblica amministrazione, quanto ad un'effettiva modernizzazione, non soltanto generazionale, ma anche infrastrutturale; le nuove tecnologie servono ad andare incontro alle richieste degli imprenditori, dei cittadini e di una società più veloce e più moderna. C'è un capitolo importante, quello della transizione energetica. Amo parlarne senza innamoramenti, perché credo che sia un obiettivo da raggiungere, se rimane una transizione sociale. Siamo la seconda seconda industria manifatturiera d'Europa e non possiamo permetterci di perdere il nostro *know-how* storico, ad esempio nel settore dell'*automotive*

energie verdi e le sostanze che possono essere utilizzate al posto della benzina per portare avanti un nuovo tipo di *automotive*, che sicuramente è più ecologico, ma non è solo elettrico. L'elettrico tal quale rischia - ahimè - di consegnare la nostra industria produttiva alla Cina. E, con tutto il rispetto per la Cina, perché fare a meno della Ferrari o di quella che un tempo si chiamava FIAT e adesso si chiamava Stellantis? Noi abbiamo le capacità

l'emendamento approvato), ma abbiamo bisogno anche di regole più semplici. È impossibile che diciamo no al nostro gas e ai rigassificatori, ma poi, quando dobbiamo fare grandi progetti di parchi eolici e di parchi solari, riusciamo a trovare comitati che dicono no anche

Noi, come Italia Viva e Azione (terzo polo), saremo sempre dalla parte del Paese e dei cittadini. Il fatto che avete colto due nostri cavalli di battaglia ci

Saremo sempre dalla parte del Paese, ovviamente con i nostri emendamenti e con le nostre proposte, che spero, come questa volta, vengano accolti con grande intelligenza e lungimiranza.

bene la collaborazione anche da parte delle minoranze, bene la disponibilità, bene il fatto che in Commissione e in quest'Aula sia chiaro a tutti che la sfida del PNRR non è dell'attuale maggioranza, ma del Paese. non ci sono dubbi ed è bene che tale idea sia consolidata in tutti noi, perché questo è il percorso che dovremo fare insieme. Va bene anche perché questa cosa è nata da una collaborazione nel lavoro all'interno della Commissione, con il Governo non si è limitato a dare pareri favorevoli agli emendamenti presentati dai colleghi della maggioranza, ma ha fatto un distinguo nel merito, come dev'essere. Va bene quindi che anche emendamenti delle minoranze siano passati, migliorando questo provvedimento. Si sapeva

con la modifica del codice degli appalti, la lentezza dell'assegnazione dei lavori per il compimento delle opere. Anche se la modifica del codice dei contratti pubblici non è ancora una risposta completa e definitiva - ne siamo consapevoli tutti - introduce però molto di ciò che serve molto di ciò che serve per smuovere il complesso pianeta delle opere pubbliche. Come ho già avuto modo di dire, in Italia la macchina complessiva degli investimenti pubblici, quando siamo bravi, riesce a investire o spendere, come meglio si vuol dire, circa 4,5 miliardi di euro l'anno. È evidente che diventa difficile pensare di moltiplicare questi investimenti per quattro o otto volte, senza radicali innovazioni. Era evidente che bisognava e temo bisognerà ancora intervenire. Credo sia necessario - è una delle poche soluzioni che abbiamo davanti - il massimo coinvolgimento del privato. Dobbiamo incentivare e sostenere il partenariato pubblico-privato, con due risultati positivi ed immediati: almeno il dimezzamento dei tempi tecnico-burocratici, mettendo a frutto la possibilità e la e la ricchezza che abbiamo nel privato nel progettare e nel portare avanti opere innovative, e l'aumento considerevole dell'importo dell'investimento, che chiaramente si riflette sul PIL e sugli effetti positivi per la nostra economia. Certamente condizione dev'essere la strategicità delle opere, in vista di una crescita del PIL e della nostra economia. del dibattito se sia meglio spendere tutto o solo una parte dei finanziamenti del PNRR, nell'incertezza della capacità d'investimento nei tempi dati, Presidente-PPE si schiera perché tutto l'investimento possibile sia messo a terra, come si usa ormai dire, ma con un'attenzione e una verifica nuove rispetto all'utilità e alla strategicità delle opere. Per queste ragioni diventano fondamentali, nel provvedimento, le misure per la *governance* del Piano nazionale di ripresa resilienza. La nuova struttura di missione PNRR, presso la Presidenza del Consiglio, sarà il punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR. bene che vengano riorganizzate le unità di missione presso le amministrazioni centrali, poste anche all'interno di direzioni generali già esistenti. Si rafforzano i poteri sostitutivi e vengono dimezzati i termini per provvedere in caso d'inerzia da parte del soggetto attuatore. Sono ipotesi che devono essere pensate e devono trovare una soluzione già da ora, perché non avremo il tempo di intervenire dopo. Allo stesso modo, sono fondamentali le disposizioni volte a favorire il controllo e il monitoraggio della spesa e degli interventi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze l'accelerazione e lo snellimento di procedure in materia di appalti pubblici e grandi opere, che, come già dicevo, rischiano di non essere sufficienti, così come recepiti nella riforma del contratto delle opere pubbliche. bene l'estensione, proprio per questo, delle procedure supersemplificate, perché ne abbiamo bisogno non solo per gli istituti penitenziari e per altre opere particolarmente importanti. per il dimezzamento dei termini per l'esproprio e per l'espressione del parere da parte della Conferenza unificata per le opere PNRR: sono tutti passaggi burocratici di cui, sì, abbiamo bisogno e non possiamo fare a meno, ma

perché non si attua il PNRR senza le imprese italiane. Non si attua il PNRR solo progettando le opere e poi lasciandole al caso. Abbiamo bisogno di imprese forti, che siano piccole, medie o grandi, ma in grado di affrontare i temi di oggi e di domani. Oggi, infatti, le nostre imprese soffrono dal punto di vista finanziario e soprattutto mancano delle dovute garanzie e della liquidità che meritano e che oggi non hanno non per colpa loro. Dobbiamo dare risposte a tutto ciò, perché la liquidità necessaria alle imprese è necessaria anche a noi e all'attuazione del PNRR, altrimenti non potrebbero operare. Da un lato, dobbiamo loro una soluzione in quanto imprese, ma, dobbiamo una soluzione anche per ciò che stiamo impostando, altrimenti il sistema non funziona e di questo dobbiamo essere pienamente consapevoli. Si è fatto tanto e questo non sarà certo l'ultimo provvedimento riguardante il PNRR,

Signora Presidente,colleghi, rappresentanti del Governo, oggi vorrei far conoscere ai cittadini in che modo la conversione in legge del decreto-legge in discussione inciderà sul loro futuro. Per far questo devo partire raccontando un fatto, o meglio le varie versioni di un fatto che rappresenta un punto cruciale per il nostro Paese. Viviamo in un Paese - e su questo non penso possano esserci dubbi - in cui abbiamo bisogno di intervenire con investimenti mai visti su sanità, istruzione, infrastrutture e via dicendo. Per diversi esponenti della Lega, però, qualcuno, sconsideratamente, al solo scopo di mettere in difficoltà il nostro Paese, ha avuto il coraggio di ottenere la fetta più consistente della cifra messa a disposizione dall'Europa per gli Stati membri per risollevare il tessuto economico e produttivo duramente colpito dalla pandemia. Si tratta di 209 miliardi. Come si è permesso Giuseppe Conte di portare tutti questi soldi in Italia? Sono troppi, spenderli Di fronte a una somma così ingente, capisco lo smarrimento del partito del ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti, che si esalta per gli appena 3 miliardi che porteranno verosimilmente un vantaggio fiscale nelle buste paga degli italiani di 8-10 euro, ben che vada; vada; nel frattempo, però, il carrello della spesa si svuota, i mutui hanno rate che salgono all'impazzata e le famiglie non riescono più a far fronte a questi impegni. Questi tre miliardi sono stati certificati ieri dal Documento di economia e finanza approvato dal Consiglio dei ministri; lo stesso documento però - ma

alle manovre espansive del secondo Governo Conte; ha certificato che non esiste nessun buco di bilancio da superbonus, altrimenti avrebbero dovuto adottare e dare evidenza a misure necessarie a coprire il fantomatico buco. Invece non c'è traccia di nulla del genere. Peccato non ci sia traccia nemmeno di uno straccio di scuse alle imprese e ai lavoratori messi in crisi dalle loro bugie. Poi ci sono quelli di Fratelli d'Italia. Questi 209 miliardi - bisogna capirli - se li sono ritrovati tra capo e collo; effettivamente, se fosse stato per loro, questi soldi non sarebbero mai arrivati in Italia, perché quelli di Fratelli d'Italia in Europa si sono astenuti ben cinque quando il Parlamento europeo ha votato sullo stanziamento di questi fondi *(Applausi),* però almeno avranno le idee chiare su come gestirli. Su questo punto però, signor Presidente, il dubbio che invece non sappiano dove mettere le mani sorge spontaneo ascoltando la Meloni dichiarare che non condivide l'allarme sollevato sui fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per i ritardi e il rischio di perderli. Tutto sotto controllo, insomma. Però, c'è un però: per il suo ministro Fitto, sodale di partito, responsabile nel suo Dicastero proprio della gestione dei fondi, è assolutamente necessario rivedere la programmazione e la riallocazione di progetti in programmi che non rischiano di perdere il finanziamento; una sfida non semplice, «da far tremare i polsi» (sto citando testualmente le parole del ministro Fitto). Ma come, la Meloni ostenta sicurezza sul polso fermo con cui il Governo sta gestendo il Piano nazionale di ripresa e resilienza e, al contempo, al suo ministro Fitto tremano i polsi?

in che modo pensa di intervenire per superare l'ostacolo incontrato dagli enti locali, per carenza di personale qualificato, nel rendere esecutivi i progetti. Accentrando forse la *governance* e rischiando di rendere più lento e farraginoso tutto il processo? domande su come pensa di riallocare i fondi in modo che i soldi vengano spesi tutti: definanziando progetti per asili, scuole, ospedali e infrastrutture, di cui il Paese ha bisogno come il pane? Questa e molte altre domande il ministro Fitto le ha scrupolosamente annotate, ma si è congedato con il più classico dei «le faremo sapere». Ancora aspettiamo. Poi non stupiamoci se alcuni amministratori locali e governatori arrembanti si sono sentiti autorizzati a fare battute infelici, per la serie: dateci i soldi che gli altri non riescono a spendere. spregio totale del vincolo di base del Piano, che ha come scopo principale quello di colmare le differenze ataviche tra Regioni di serie A e Regioni di serie B, tra i centri ricchi e le periferie povere in tutto il nostro Paese. rappresentanti del Governo, diciamolo agli italiani: l'Italia qui si gioca il proprio futuro; si gioca la possibilità del più grande rilancio e ammodernamento di tutti quei settori in cui siamo da sempre il fanalino di coda in Europa, la cenerentola dei Paesi più avanzati dell'Occidente. Ci giochiamo il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti, e non possiamo sbagliare. Nella maggioranza e nel Governo in molti siedono tra questi banchi da più di trent'anni. Sono molto preoccupata, signor Presidente, perché trent'anni fa sui libri universitari leggevo della questione meridionale, che già allora era un'emergenza *(Applausi),* che costringeva molti a lasciare le periferie e le città più povere per cercare fortuna nei centri più ricchi. Leggevo di scelte della politica che avrebbero pesato sulle generazioni future. Immaginate cosa ho pensato e provato quando ho compreso di essere io quella generazione futura. Poi non stupiamoci se le persone e i giovani non credono più nella politica e non vanno più a votare. Per far tornare le persone a votare non serve certo abbassare al 40 per cento la soglia per l'elezione diretta dei sindaci, come la maggioranza ha già tentato subdolamente di fare con emendamenti presentati alla chetichella. Il motivo per cui abbiamo registrato tassi *record* di astensione è che le persone che vivono tutti i giorni sulla pelle inefficienze e diseguaglianze, in trent'anni non hanno ricevuto risposte. In questo Governo, invece, si è mantenuta la pessima abitudine di scaricare i fallimenti della della politica sui giovani. Purtroppo lo sanno bene i giovani fuori da quest'Aula, che si sentono dire, da quando questo Governo si è insediato, che devono smettere di inseguire i loro sogni e accettare la prima offerta di lavoro che arriva loro, anche se sottopagata e con turni massacranti. L'aggravante è che questa gavetta, che in questo caso diventa sinonimo di sfruttamento, poi non si concretizzerà in un lavoro soddisfacente in futuro. Infatti, con il ripristino dei *voucher* e l'innalzamento del tetto delle prestazioni occasionali a 10.000 euro, spingete i giovani in un'unica direzione, quella del precariato selvaggio. Purtroppo lo sanno bene anche gli imprenditori, ai quali, per puro furore ideologico, avete tolto uno strumento come Transizione 4.0, l'unica misura che in questi ultimi anni ha consentito loro di ammodernare i mezzi e far crescere professionalmente la forza lavoro senza pesare sulle casse delle imprese. E menomale che almeno non avete tolto e avete mantenuto gli sgravi introdotti dal governo Conte II con decontribuzione Sud, misura che avete avuto l'impudicizia di appuntarvi al petto, propagandandola come fosse una vostra medaglia. Ma siamo seri! Comprenderete quindi, Presidente, colleghi, quanto grande possa essere il timore per questa manifesta incapacità del Governo di fornire prima di tutto ai cittadini risposte serie e trasparenti sull'andamento della gestione di questi 209 miliardi. Ricordo a me stessa e a tutti noi che il Governo è in carica ormai quasi da sei mesi e anche i cittadini che hanno dato fiducia a chi si è detto pronto iniziano a chiedersi quando arriveranno le prime soluzioni concrete da parte di Giorgia Meloni e dei suoi Ministri. In conclusione, qualunque sia la versione che questa maggioranza prova a dare di come sono arrivati e di come si devono gestire i 209 miliardi, dev'esserci un unico finale possibile: questi soldi li dobbiamo spendere tutti e li dobbiamo spendere bene. Ne abbiamo assolutamente bisogno. Per questo, come opposizione responsabile, ci siamo messi a disposizione per dare il nostro contributo costruttivo e fattivo. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza è l'ultimo treno per un futuro di sviluppo e rilancio dell'Italia e non c'è spazio per sacrificare nemmeno un centesimo per propaganda elettorale o per appagare appetiti di parte. Ricordiamo - e concludo, Presidente - che l'Italia tutta ha ottenuto questi 209 miliardi anche per il prezzo pagato in vite umane durante il periodo più nero che abbiamo attraversato nella storia più recente. Anche per loro, per quelle vite spezzate, abbiamo il dovere di centrare tutti gli obiettivi: fallirne anche solo uno non è un'opzione contemplabile.

che abbiamo in discussione in questo momento introduce misure per il rafforzamento delle amministrazioni che sono coinvolte nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e consente anche di riorganizzare le strutture preposte al coordinamento della gestione, al monitoraggio, alla rendicontazione e al controllo del Piano. Si tratta quindi di un provvedimento di grande importanza, che agisce sulla stessa attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, misura fondamentale, che darà al nostro Paese il sostegno e la spinta necessaria alla ripresa e all'innovazione, se potrà essere attuata in tempi brevi. Mi permetto di ricordare che l'Italia è il principale beneficiario del fondo del Next generation EU. La maggior parte dei Paesi ha fatto domanda solo per la parte di risorse erogate sotto forma di sovvenzioni e solo sette Paesi hanno richiesto anche i prestiti. L'Italia si colloca in prima posizione, ma, a prescindere da questo, il disegno di legge include misure importanti anche per quanto riguarda il Dicastero delle imprese. Il provvedimento interviene sulla disciplina che consente l'utilizzo dell'ammontare dei finanziamenti garantiti da SACE per le imprese energivore, colpite dagli effetti negativi del conflitto russo-ucraino, ai fini della copertura del fabbisogno di liquidità delle medesime imprese (per i successivi dodici mesi, se piccole e medie imprese, oppure sei mesi, se grandi imprese). Nella direzione delle modifiche apportate in Commissione va anche l'emendamento che ho presentato insieme alla collega Murelli e ad altri colleghi della Lega, approvato in Commissione bilancio, che prevede l'estensione del programma di massimizzazione previsto per gli impianti alimentati da biomassa liquida anche a quelli di biomassa solida per garantirne la continuità produttiva. Nel nostro Paese numerose centrali a biomassa legnosa hanno interrotto la produzione, compromettendo la tenuta dell'intero settore con impatti importantissimi sull'occupazione. Questa misura non solo interviene in tema di energia, ma serve anche a tutelare le foreste, i boschi e l'ambiente. Da tempo le imprese boschive ci segnalano l'esigenza di provvedimenti tempestivi volti a sostenere la produzione delle centrali con benefici per l'intera filiera del legno. L'assenza poi di un monitoraggio costante delle risorse forestali alimenta il rischio concreto di incendi e di calamità che le attività di silvicoltura contribuiscono a scongiurare, favorendo la stabilizzazione del suolo ed evitando la perdita di milioni di ettari di risorse boschive. Negli ambiti degli stessi interventi per la tutela del territorio e della risorsa idrica, tra gli emendamenti approvati ce n'è anche uno nostro nel quale siamo riusciti a prorogare il termine di completamento delle sperimentazioni sul deflusso ecologico, la cui entrata in vigore viene posticipata al 30 giugno 2025. Non è banale questo emendamento, ma è molto importante, perché questa misura, in un Paese oggi a rischio siccità in aree molto ampie, diventa fondamentale per la tutela della risorsa idrica, ma soprattutto per il suo utilizzo da parte di coloro che svolgono attività agricola. Le sperimentazioni previste per l'entrata in vigore del deflusso ecologico non sono attuabili, se non

L'emendamento, riformulato dal Governo, prevede che non ci sia alcun compenso aggiuntivo per il commissario, che potrà agire rapidamente, perché avrà a disposizione un progetto definitivo e finanziato. Come ha sottolineato il sindaco della città di Torino,

risposte concrete a un *dossier* importantissimo sulla città capoluogo di Torino, ma che coinvolge l'intera Regione Piemonte. La *governance* - signor Ministro, lo dico a lei, ma anche al al Presidente dell'Assemblea - passa necessariamente attraverso le persone che devono attuare le norme e gli investimenti. Su questo tema il Governo ha cercato di indirizzare tutti i suoi sforzi e bene ha fatto, perché ci dimentichiamo sempre delle persone che poi devono fare le cose. Noi trattiamo sempre l'argomento del Piano nazionale di ripresa resilienza con una visione economica e numerica: ma chi deve attuarlo sono donne e uomini come noi, che hanno bisogno di sostegno e di fiducia anche da quest'Assemblea e ciò diventa fondamentale. *(Applausi)*. A tale proposito voglio citare una frase importante, non di un pericoloso sovranista, ma di una persona straordinaria, immensa, di fede e di pace come Papa Francesco: «L'uomo non è un fattore economico in più, o un bene scartabile, ma qualcosa che ha una natura e una dignità non riducibili a semplici calcoli economici». A mio parere, questa è l'ispirazione che ci deve portare avanti, soprattutto quando prendiamo decisioni importanti, che hanno effetti su questi provvedimenti, che sono stati oggetto di critica politica da parte di più Gruppi, ma, dall'altra parte, avranno un effettivo valore se riusciremo ad attuarli in tempi brevi e, soprattutto, con la massima concretezza, come si addice a questa maggioranza politica. Grazie, signor Ministro. Grazie, Presidente.

invece, di alcuni temi, che soltanto in parte sono stati sfiorati da un dibattito sicuramente interessante, che il Partito Democratico ha affrontato con spirito costruttivo, ma che, dopo tre ore in quest'Aula, mi lascia un po' perplessa.

se abbiamo fatto bene o male come sistema Italia ad accettare e a volere circa 200 miliardi di investimenti e di prestito europeo per rilanciare la nostra Nazione e la nostra economia, ma soprattutto intervenire sui sei pilastri che riteniamo necessari per affrontare - con la giusta cassetta degli attrezzi - le sfide del futuro, tra cui la digitalizzazione, l'energia, l'ambiente e la sanità.

l'Italia non è in grado normalmente di spendere i fondi strutturali, e cioè le risorse assegnate. Credo che questo sia un punto di partenza oggettivamente perdente

un Paese si misura anche sulla sua capacità di spendere quello che chiede e di portare a casa gli investimenti per cui ha lottato, e portare a casa 200 miliardi di investimenti, anche nella parte a prestito, è a mio avviso avviso essenziale - ed esiziale - per il nostro futuro, per lo sviluppo, per il PIL e per la crescita dell'Italia, soprattutto se lo mettiamo a confronto con l'altro dato di oggi, e cioè la presentazione del Documento di economia e finanza, il DEF, in cui si traccia una strada non certamente brillante per il Paese sia sull'impatto del PIL sia per quanto riguarda quelli che dovrebbero essere i finanziamenti strutturali del nostro Paese, tra cui quelli sulla scuola e sulla sanità. Quando parliamo di PIL, vorrei ricordare che il PNRR, che non è un fondo di coesione, ma si basa sulla capacità di *performance* del Paese - quindi è una scommessa sulla nostra capacità di sviluppo e di crescita - incide, a base normale al 2026, per l'1,9 del PIL come impatto e al 2036 per il 13 per cento. È cioè un elemento di volano e di sviluppo della nostra economia che difficilmente potremmo immaginare di avere. Uno degli aspetti principali di cui non si è discusso in questo questo dibattito è non solo come mettere a terra i progetti, ma anche le riforme necessarie, che continuiamo a presentare in questo nostro Parlamento con finanziamento pari a zero, cioè, con copertura zero, come abbiamo fatto recentemente sulla riforma sociosanitaria.

non è la riforma Calderoli, non è quella. Nella maggioranza abbiamo due ragionamenti diversi e ad oggi

In questo contesto permettetemi però di dedicare alcuni minuti al tema sanitario: la sanità è uno dei pilastri del PNRR, la sesta missione, ma non è un pilastro che si fa da solo. Poco ne abbiamo parlato durante questo dibattito ed erano pochi gli emendamenti presentati. È un

e dei tagli del passato, ma qual è la quotidianità che vediamo oggi? Sono i tagli del presente. Il DEF che ci è stato presentato ieri, o almeno di cui abbiamo letto sulla stampa, di fatto congela la situazione del bilancio del bilancio degli scorsi anni, cioè quella del 2023-2025, con un tendenziale del Fondo sanitario che scende, in termini percentuali cento. La questione essenziale è: il Fondo sanitario nazionale aumenterà nei prossimi anni o diminuirà? Il Fondo diminuisce e, se diminuisce, non serviranno certo gli 1,1 miliardi che abbiamo avuto nel decreto bollette per risolvere i problemi di oggi e cioè la mancanza strutturale e strutturata di personale sanitario, di politiche economiche sanitarie per l'assunzione, la formazione e l'adeguamento del personale sanitario, senza la quale il sesto pilastro del PNRR, cioè la parte relativa alle Case della comunità e all'adeguamento della medicina territoriale, la famosa medicina del territorio, non si può fare

che l'*austerity* dovrebbe essere finita e questo lo dice chi l'*austerity* l'ha subita. Se l'*austerity* è finita dobbiamo fare delle scelte; le scelte si finanziano e uno dei pilastri di queste scelte è garantire la sicurezza del Servizio sanitario nazionale pubblico nel nostro Paese.

e neanche in questa occasione di semplificazione normativa e di messa in campo non abbiamo risposte. Non sappiamo, Ministro, se questi 100 miliardi li perdiamo o no. Spero che oggi sia la volta buona e che qualcuno, in sede di replica, ci dica chiaramente se questi 100 miliardi del PNRR noi li perdiamo. Faremo

di diagnosi, che sia a Bolzano o a Reggio Calabria, dovrebbe essere lo Stato organizzato a pagare. Lasciamo stare i Governi; voi vi siete storicamente occupati più di privato accreditato che di sanità pubblica. *(Commenti*.

Purtroppo, la mia Regione ha un ritardo strutturale maggiore. Qual è la grande difficoltà per cui penso che il dibattito vada inquadrato nella visione politica di un nuovo Governo? Non c'è soltanto

Regione. Il Mezzogiorno ha un ritardo strutturale antropologico, ma anche un ritardo strutturale patriottico, perché per quanto mi riguarda ogni punto di PIL in più nel Veneto o nella Lombardia è una grande opportunità anche per chi vive nel Mezzogiorno. Oggi venivo da una visita al Gemelli dove la maggior parte dei primari sono calabresi, mentre al Sud c'è una disoccupazione intellettuale

un'Europa della sfida: si dibatte tanto su quanta autonomia debba esserci in questa sfida, perché abbiamo una guerra alle porte, rispetto al tema della Cina, rispetto al tema di una Russia che

Signora Presidente, ringrazio tutti i colleghi che sono intervenuti in questo dibattito. Voglio rivolgere un ringraziamento innanzitutto al collega Calandrini, ai colleghi Testor e Gelmetti, come relatori di questo provvedimento, e a tutti i membri della Commissione, perché ritengo che si sia riusciti a fare un ottimo lavoro in Commissione, che è stato un po' tradito - devo dire - dallo spirito di questo dibattito. Mi sia consentita questa premessa, perché quello che è accaduto in Commissione non è quello che è accaduto in Aula. Comprendo le ragioni della politica, perché ho iniziato da qualche giorno ad avere questo impegno, però chiaramente è necessario sottolineare tutto questo lavoro, perché ritengo che altrimenti rischieremmo di parlare di altro e non invece del merito del provvedimento. Ritengo che sia molto utile, invece, fare alcune riflessioni sulle questioni di merito del decreto-legge, il quale si inserisce non in un'occasione di scontro e di polemica, ma in una visione che questo Governo ha avuto sin dal primo momento e che noi rivendichiamo con forza e con decisione. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri ha ritenuto di individuare, nella scelta dell'accorpamento di alcune deleghe, una linea di marcia e di tendenza, ha già compiuto una scelta che ha una visione e che indica la complessità delle questioni di fronte alle quali ci troviamo. Nel momento in cui si è deciso di mettere insieme il Piano nazionale di ripresa e resilienza con la politica di coesione, si è fatta già una scelta *(Applausi)*, una scelta importante che parla a un grande problema di questo Paese. È inevitabile, per avere l'approccio giusto all'analisi del decreto-legge, fare anche alcune riflessioni di merito, perché, se in questo decreto abbiamo sostanzialmente tre questioni insieme, non si tratta della somma di cose diverse, ma dell'inizio di un percorso di coordinamento su questa strategia. C'è un tema che affronta la *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza,

proprio perché le due questioni non possono essere scollegate, come si rischiava di fare. È importante anche su questo fare una premessa, che non è casuale.

mesi, meno di sei, lo dico per inquadrare la discussione rispetto a un elenco di questioni sulle quali tornerò e rispetto anche alle sollecitazioni che ci sono state. Eppure il Governo ha compiuto la prima scelta di andare a verificare, con una relazione precisa e puntuale, lo stato di attuazione delle politiche di coesione nel nostro Paese, perché, a furia di parlare solo di PNRR, si perdono dei punti di riferimento essenziali per capire come poter utilizzare queste risorse e soprattutto per capire quale può essere la proiezione futura che vada oltre il Piano nazionale di ripresa di residenza.

evidenzia una seconda questione collegata non alla relazione di cui abbiamo discusso e su cui torneremo, rispetto al decreto della Corte dei conti, ma a quella precedente relativa all'analisi dell'uso di queste risorse. risorse. Un terzo punto di riferimento sono i dati della Ragioneria generale dello Stato sull'uso delle risorse della programmazione 2014-2020. Pensiamo di non doverne parlare? Pensiamo di dover parlare immediatamente di quello che succederà? O vogliamo partire invece da questa diagnosi, per immaginare - mi auguro insieme, perché il tema non è di parte - una terapia utile per dare al nostro Paese delle soluzioni reali e credibili? Di questo noi parliamo. Allora bastano - ahinoi - pochi numeri per fotografare questa situazione, perché nella programmazione 2014-2020, a fronte di 126 miliardi di di euro assegnati al nostro Paese, tra risorse europee, risorse nazionali di cofinanziamento, risorse regionali e risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), i dati ci indicano che, a due mesi fa, la percentuale di spesa è pari al 34,5 Questo è un dato. Vogliamo far finta che non ci sia? A fronte di 126 miliardi di euro, nel 2023, dopo nove anni, circa di spesa. Ma qui le giustificazioni sono tante. Noi abbiamo speso i soldi europei? Sì, perché la composizione di questa articolata questione pone insieme le risorse dirette europee, il cofinanziamento nazionale, il cofinanziamento regionale e mette insieme il Fondo per lo sviluppo e la coesione. È evidente che se mettiamo da parte tutti quei fondi che non devono essere rendicontati, ci concentriamo esclusivamente sulla parte europea e ricordiamo - perché è giusto farlo - che da quei fondi sono state prelevate le risorse per affrontare l'emergenza pandemica, con il loro utilizzo per

perché è evidente che oggi siamo in una fase nella quale, nei mesi prossimi, da qui al 31 dicembre 2023, dovremo completare la programmazione della coesione, per la parte delle risorse europee ancora da spendere, dovremo essere - e lo siamo: poi tornerò nel merito - in piena corsa sull'utilizzo delle risorse del PNRR e dovremo iniziare a spendere le risorse della programmazione di coesione 2021-2027, che sono oltre 40 miliardi di euro di risorse europee, più il cofinanziamento, l'FSC e tutto quello che ci porta ad una dimensione del problema che è leggermente più grande della semplificazione che ho ascoltato oggi, rispetto a chi deve spendere e chi deve invece dire come si spendono le risorse. *(Applausi)*. Il richiamo che faccio è al clima emerso nei lavori di Commissione, perché in Commissione questa consapevolezza, presidente Calandrini, è emersa. Lo sanno i relatori e lo sanno tutti i colleghi che hanno lavorato. Purtroppo qui in Assemblea questo si è perso e mi dispiace, perché è prevalsa - lo ripeto - la posizione politica e ne prendo atto,

approvato. Allo stesso modo abbiamo approvato numerosi emendamenti proposti dal Partito Democratico e dal Gruppo MoVimento 5 Stelle. È vero o non è vero che in Commissione abbiamo dato parere favorevole e abbiamo approvato numerosi emendamenti proposti dagli altri Gruppi?

con qualche collega se entro nel merito del provvedimento di cui stiamo parlando, perché ho sentito tante cose un po' fuori tema rispetto al merito del provvedimento. *(Applausi)*.

sono state delle proposte e dei suggerimenti. Sapete com'è finita? Lo dico a molti colleghi che hanno detto che ci sono i Comuni e le Regioni sul piede di guerra nei confronti di questo decreto-legge, perché staremmo sfasciando tutta la gestione perfetta che c'era. Ebbene, in sede di Conferenza unificata,

guardato al merito del provvedimento e hanno dato risposte positive, perché il confronto è stato utile. Non è un caso che dentro questo decreto ci sia una parte centrale molto importante che affronta il tema delle semplificazioni e delle accelerazioni, in cui abbiamo recepito molti suggerimenti e indicazioni che sono venuti dal sistema delle autonomie locali, perché essendo impegnati direttamente in trincea hanno posto alcune questioni, che erano state poste molte volte e molto tempo prima e che ora sono state accolte. Non è tutto? È poco? Non lo so. Io dico che intanto si è compiuto un primo passo molto importante in questa direzione, perché sono stati recepiti questi emendamenti e sono stati portati all'interno di un testo che è migliorato e che ha due aspetti altrettanto importanti quando parliamo di *governance* sia del PNRR che della coesione. Ho ascoltato molte cose che mi limito a definire inesatte,

faccio alcuni esempi concreti per rimettere ordine anche nella verità delle cose, nei processi ai quali si è fatto riferimento - abbiamo recepito alcune indicazioni della Corte dei conti

che in due anni, così come la Corte dei conti indica in modo molto chiaro, quelle strutture, che erano nate nei Ministeri per avere una professionalità e una competenza finalizzata a gestire una fase complessa per tutto il periodo dell'attuazione del PNRR, invece andavano smantellandosi perché, siccome c'erano rapporti di collaborazione a tempo determinato, molte di queste persone trovavano molto più utile andare presso altre amministrazioni, in altre situazioni. Pertanto, quando abbiamo messo mano alla questione, abbiamo verificato che

di opinioni; metto sul tavolo le questioni vere, reali, sulle quali noi ci confrontiamo ogni giorno rispetto alle difficoltà che ci sono nella gestione di una situazione così complessa. Quando si parla del rapporto di contrapposizione tra MEF e Presidenza del Consiglio si dice un'altra inesattezza. Questo Governo ha fatto la scelta di mettere in campo un Ministero per l'attuazione del programma. C'è qualcuno che può contestare il fatto che ci sia l'esigenza di avere un luogo di coordinamento nell'attuazione di un programma da 220 miliardi di euro, oppure dovevamo immaginare che questo potesse andare avanti con le modalità precedenti? Vogliamo parlare nel merito delle diverse istituzioni, dei diversi uffici, delle diverse segreterie e di tutta una situazione interna nelle diverse amministrazioni dello Stato, avendo la necessità e l'obbligo di distinguere i ruoli e le funzioni? Vi è, infatti, chi si occupa dell'attuazione di alcune misure e c'è chi deve coordinare e monitorare l'attuazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze mantiene tutta la parte relativa al monitoraggio e all'attuazione - e ci mancherebbe altro - della parte finanziaria del programma e provvede anche all'inoltro delle richieste di rate di finanziamento da parte della Commissione europea.

Abbiamo anche compiuto un'altra scelta che rivendichiamo: avevamo due nuclei rispettivamente di 30 e 32 persone; li abbiamo soppressi e ne abbiamo creato uno solo di 40 persone riducendo la spesa, perché - e lo voglio sottolineare con forza - si può riorganizzare si può riorganizzare senza necessariamente assumere ed aumentare le spese. Questo decreto-legge riorganizza e potenzia le strutture dei luoghi nei quali è necessario potenziarle, ma costa molto meno di quanto costavano le precedenti strutture *(Applausi)*,

delle semplificazioni, alcune trasversali, ed alcune tematiche che hanno affrontato nodi e questioni che esistevano da tempo. Troverete all'interno del provvedimento anche alcune scelte che hanno affrontato e risolto, sul fronte della semplificazione e dell'accelerazione, situazioni annose che rischiavano di compromettere l'avanzamento del PNRR. Non lo diciamo noi; ce le hanno chieste i Comuni, le Regioni, le Province, i vari interlocutori, e noi le abbiamo accolte ed inserite, proprio per avere l'obiettivo opposto a quello che ci viene rimproverato, ossia una accelerazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Detto ciò, rispetto alle questioni sollevate durante il dibattito, alcuni chiarimenti sono d'obbligo. A me dispiace che alcuni parlamentari e alcune senatrici che sono stati prodighi di suggerimenti e di critiche adesso non siano qui in Aula. Ho ascoltato con doverosa attenzione tutto il dibattito *(Applausi)* e mi sarei aspettato che, in sede di replica, fossero presenti anche questi interlocutori, anche e soprattutto per poter chiarire alcune inesattezze ulteriori. La prima inesattezza è collegata al codice degli appalti. Peccato che ci sia una clausola nel codice degli appalti che il ministro Salvini, tanto criticato, ha inserito e che prevede, d'accordo con la Commissione europea, la sua non applicazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Quindi è un problema che raccontiamo ma che non corrisponde alla realtà dei fatti, perché non produce quegli effetti così disastrosi ai quali si fa riferimento. Peccato che il codice degli appalti, precedentemente e non da noi, è stato individuato come uno degli obiettivi al 30 marzo, quindi andava approvato in Consiglio dei ministri entro tale data. L'entrata in vigore avverrà il 1° luglio e sarà oggetto di un confronto con la Commissione europea per valutare insieme se una riforma così sostanziosa è utile che parta subito o è necessario che tenga conto anche della fase nella quale ci troviamo, rispetto all'avvio di questi investimenti. A me non piace partecipare A me non piace partecipare al dibattito a proposito di chi sia il merito, perché la polemica è fine a se stessa, ma suggerisco la lettura del

Si parla sostanzialmente di tre criteri: uno è quello del maggior calo del PIL nel periodo della pandemia; il secondo è quello della crescita della disoccupazione; il terzo è quello del numero degli abitanti in rapporto alla popolazione europea. Sono dati che, con tutto lo sforzo che possiamo fare, mi mettono in difficoltà nell'attribuire dei meriti obiettivamente rispetto all'ottenimento di queste risorse. *(Applausi)*. Il tema è un Il tema è un altro, ma ne parleremo successivamente, perché con piacere sarò presente in Parlamento per l'informativa richiesta e con altrettanto piacere, subito dopo, avremo un dibattito sulla relazione semestrale, nella quale fotograferemo nel suo insieme la dimensione, le criticità, i problemi, le scelte e le soluzioni rispetto al Piano nazionale di ripresa resilienza, facendo quindi quello che stanno facendo tutti gli altri Paesi europei. Solo che in Italia questo è diventato un dibattito con il quale in ogni circostanza si immagina di poter colpire o criticare questa o quella dichiarazione. Ma a me sembra che la situazione di fronte alla quale ci troviamo sia diametralmente opposta a quella che in alcuni casi viene rappresentata. Ciò perché è evidente che ci sono dei dati oggettivi che vanno ricordati. Il primo: il Piano nazionale di ripresa e resilienza è stato deciso prima dello scoppio della guerra, prima dell'invasione da parte della Russia dell'Ucraina. Mi sembra che ci sia un dato oggettivo sul quale riflettere. Il primo dato è che in un Piano che prevede circa 110 miliardi di euro per opere pubbliche, il tema dell'aumento del costo delle materie prime in qualche modo inciderà. È questo un primo tema che non decide questo o quel Ministro, questo o quel Governo, ma è un dato oggettivo. La seconda questione, altrettanto collegata, è che cambiano le priorità rispetto a quella programmazione. Non è un caso che nel RRF, l'articolo 21 stabilisce che in caso straordinario si possa immaginare una modifica del Piano. Ritengo che chi ha scritto quell'articolo 21 mai potesse immaginare in quel momento una guerra; mai potesse immaginare in quel momento che la causa straordinaria potesse essere una guerra così vicina ai nostri confini. Questi sono però, consentitemi, dati oggettivi, che aggiungo anche con un collegamento alla coesione. Infatti anche l'accordo di partenariato, lo strumento europeo che approva i programmi italiani sull'utilizzo della politica di coesione per il 2021-2027,

C'è l'esigenza di una riflessione a 360 gradi per capire come rendere attuali questi interventi? E, soprattutto, se l'Italia ha 48 programmi all'interno della politica di coesione e primeggia, per questo sì, rispetto agli altri Paesi, c'è il rischio che l'utilizzo di queste risorse non vadano nella finalizzazione opportuna che è quella di una concentrazione auspicabile per dare una risposta strategica alle grandi questioni del nostro Paese? Noi riteniamo di sì ed è questo uno dei temi sui quali è importante ragionare.

per alcuni versi, perché indica una direzione di marcia fondamentale per modificare alcune situazioni in settori fondamentali della vita economica e sociale del nostro Paese. È però anche un tema che ci deve portare a riflettere rispetto alla tempistica dell'attuazione di queste riforme ed anche

la tempistica non è un dettaglio, ma rischia di essere devastante rispetto ad altre situazioni, è un aspetto importante sul quale lavorare d'intesa con quello che ci dicono tutti i principali attori del sistema economico del nostro Paese in questa direzione. Qui si gioca la partita delle scelte che dobbiamo fare.

diverse e numerose occasioni di confronto in Parlamento perché penso che sia doveroso farlo, anche per riportare i contenuti e gli avanzamenti di tutto quello che stiamo facendo. Consentitemi

l'approccio non è quello volto a costruire polemiche e scontri. L'approccio è differente ed è politico solamente su questo punto. Noi, per la prima volta, ci troviamo di fronte a un Governo che non deve guardare alla scadenza degli obiettivi del del 30 marzo, di giugno, del 31 dicembre di un anno senza avere l'orizzonte temporale successivo; questo Governo ha in mente il giugno 2026 perché l'orizzonte temporale è la legislatura *(Applausi)*. Quindi noi oggi abbiamo il dovere di capire quello che può essere un rischio per evitare una inutile baruffa, che magari fra uno o due anni può avvenire su chi dovesse avere la responsabilità di questo o quel mancato intervento. Capiamo adesso se alcuni di questi interventi non possono essere realizzati. E su questo ci viene incontro, anche qui, non l'opinione del Ministro o del Governo, ma la proposta della Commissione europea perché, nel momento in cui la Commissione europea approva il REPowerEU, sta dando un'indicazione di marcia, corregge il tiro, capisce che con la guerra è accaduto qualcosa che può essere la sponda per l'articolo 21. La stessa Commissione europea ci dice

aziende di Stato rispetto agli interventi da realizzare sul fronte infrastrutturale. C'è poi anche una delle questioni che è stata oggetto della discussione in Commissione e che sarà oggetto anche degli ordini del giorno, vale a dire come il REPower possa parlare anche dal punto di vista degli incentivi per l'efficientamento energetico a famiglie e imprese, non con interventi di urgenza, com'è stato fatto fino a oggi, anche utilizzando le risorse REACT-EU, ma con interventi di merito, che possono essere strutturalmente in grado di ridurre la capacità di consumo, mettendo in campo quindi una strategia differente. Il REPower sarà un capitolo aggiuntivo e questo è un passaggio altrettanto importante, che vorrei sottolineare, non dico per correggere alcune inesattezze, ma per acquisirlo come consapevolezza generale. Il REPower italiano, a differenza di quello degli altri Paesi, non avrà una grande fonte di finanziamento perché l'Italia, come tutti avete ricordato parlando di 220 miliardi, ha preso 68 miliardi a fondo perduto, 122 a debito e 30 di fondo complementare di risorse nazionali: questa è la composizione del nostro Piano nazionale di ripresa e resilienza. All'interno di questa composizione esiste la parte relativa alla quota a debito, che ha visto l'Italia prendere al 100 per cento l'intera sua quota

ci sono Paesi che stanno discutendo se, come e per cosa prendere le risorse a debito sul fronte degli investimenti; noi, invece, dobbiamo articolare il nostro REPower su due fonti di finanziamento che la Commissione europea ci indica: la prima è quella collegata a 2,7 miliardi di fondi di fondi ETS per le missioni che vengono assegnati automaticamente al nostro Paese; la seconda è quella fino al 7,5 per cento della politica di coesione. Ce lo dice la Commissione europea, non lo diciamo noi. Dunque, aver messo insieme PNRR e coesione, immaginare dei vasi comunicanti fra questi due programmi è un punto centrale che fa parte della possibilità di finanziare il REPower, che avrebbe da questa fonte di finanziamento circa 3 miliardi di euro, probabilmente non sufficienti. L'idea quindi, se vogliamo mettere in campo un REPower serio e credibile, è quella di costruire uno strumento che sia in grado di utilizzare parte di quelle risorse, laddove dovessimo accertare che quelle risorse non troveranno un completamento di spesa nel PNRR a giugno 2026. Oppure vogliamo aspettare di assistere al fatto che queste risorse non saranno spese rispetto a dei dati oggettivi? Per evitare di definanziare degli interventi - così sveliamo anche quest'altro arcano, che rischia di generare una polemica - la nostra proposta, della quale siamo convinti, è che proprio perché

giugno 2026 con il PNRR, anziché perderne l'avvio, la fase di progettazione e di gara, possono essere spostati su un fondo, quello della coesione, che ha il 31 dicembre 2029 come data di rendicontazione finale. A questo si aggiunge il tema del Fondo per lo sviluppo e la coesione, che è il terzo fondo che completa il quadro, in una visione strategica globale che il Governo mette in campo per poter dare una soluzione a tutti i problemi, affrontando queste difficoltà. che sarà oggetto di un confronto - e lo è già - con la Commissione europea: ho incontrato numerose volte i commissari europei, la *task force* e i tecnici della Commissione europea, per cui stiamo lavorando su queste ipotesi. E quando questo quadro sarà sarà predisposto, sarà portato all'attenzione del Parlamento, ci mancherebbe altro perché, così come abbiamo fatto sulla politica di coesione - non c'era nessun obbligo, è stata una scelta - faremo su tutto il resto. Riteniamo infatti fondamentale mettere in campo una capacità di azione mirata e finalizzata all'ottenimento di un risultato complessivamente positivo per il Paese, dandoci la possibilità di utilizzare, sì, tutte le risorse - e non c'è discussione su questo - ma di farlo in modo anche efficace ed efficiente. Il tema, come è stato detto, non è solamente la quantità della spesa, che pure è importante; c'è anche un tema di qualità della spesa, perché quando ci indebitiamo, stiamo pesando sul futuro delle nostre generazioni, sui nostri figli. Abbiamo quindi il dovere di immaginare che quel debito sia per interventi realmente utili e positivi per il nostro Paese. *(Applausi)*. È questo il tema che viene posto nel dibattito politico che stiamo cercando di portare avanti.

perché sarebbe anzitutto ridicolo, e poi paradossale; quindi, da parte nostra non ci può essere, in alcun modo, un'accettazione di questo tipo di impostazione. immaginiamo e che portiamo a quest'Assemblea è che si apra un confronto serio, nel merito, e che su questo confronto ci possa essere la capacità non di critiche di carattere generico, ma di proposte concrete sulle quali poter dare risposte. Faccio un'ulteriore riflessione che era sfuggita e che è importante, per dare anche l'idea - lo dico alla senatrice Lorenzin - della metodologia, di quello che dobbiamo evitare che accada e di quello che dobbiamo correggere. Avere inserito gli ospedali di comunità

che, su diversi settori del Piano nazionale di ripresa e resilienza, crea potenzialmente dei problemi. È evidente che in questo senso c'è la storia di interventi, che è stata anche richiamata nel dibattito, che ci viene incontro. Il nostro auspicio - e concludo veramente - è che su questi temi ci sia realmente un approccio serio e costruttivo, che noi siamo convinti di volere e dover recepire; ma le parole d'ordine sono serietà e responsabilità. Diversamente, c'è una polemica politica che non serve a nessuno.

Signor Presidente, colleghi, oggi alle 15 c'è stato l'ultimo saluto ad Andrea Papi: un ragazzo di soli ventisei anni amante della natura, dello sport e della montagna; un ragazzo nel pieno della vita, con tanti sogni da realizzare. Una famiglia, una comunità e tutta la gente di montagna oggi piangono un loro figlio: Andrea, di cui in questi giorni tutti abbiamo sentito parlare per la sua tragica morte, per quell'incontro con l'orso che ha spento il suo sorriso, e mi stringo a tutta la sua famiglia e alla comunità in questo doloroso momento. Quello che è avvenuto a Caldes è il tragico epilogo di tanti allarmi lanciati dal territorio, dalle istituzioni locali e dai parlamentari, rimasti inascoltati nel corso degli anni. Il progetto Life Ursus aveva previsto la reintroduzione di una cinquantina di orsi sulla base di un ampio arenale di distribuzione, che doveva andare oltre i confini del Trentino, ma che ha portato alla situazione attuale di oltre cento esemplari concentrati in una zona piuttosto ristretta, generando una forte densità di individui stanziali in un'area fortemente antropizzata. La Provincia di Trento aveva chiesto di poter intervenire con urgenza nei confronti dei grandi carnivori problematici e sottolineato la necessità di realizzare al più presto un piano di contenimento degli orsi, visto il numero diventato ormai eccessivo rispetto alla morfologia del territorio. Tale situazione rende di fatto sempre più difficile il rapporto con il nostro territorio da parte di cittadini e turisti, che si sentono sempre più minacciati, incidendo sempre più sul fenomeno dello spopolamento delle zone di montagna e sull'abbandono dei pascoli dell'alpeggio, traducendosi quindi in una riduzione della cura del territorio. Da tempo le Regioni attendono un piano di gestione dei grandi carnivori da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza con il supporto di ISPRA, per cui ringrazio il ministro Pichetto Frattin per l'incontro avuto ieri col presidente Fugatti, che auspico porti ad una soluzione del problema, con l'auspicio che ISPRA metta da parte la posizione rigida e ideologica intrapresa fino ad oggi e che si dia seguito alle richieste delle Regioni

Abbiamo presentato come parlamentari, sia al Senato che alla Camera, un disegno di legge che assegna la gestione dei grandi carnivori alle Province autonome e alle Regioni. questo tragico episodio, che il disegno di legge venga incardinato. Noi vogliamo che questo ragazzo ritrovi la sua dignità e che questa famiglia trovi risposta in azioni concrete. Basta ideologie: lo dobbiamo ad Andrea, lo dobbiamo alla sua famiglia, lo dobbiamo alla comunità, lo dobbiamo alla gente di montagna. *(Applausi)*.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 Comunico che, in accordo con la Presidenza della Camera dei deputati, le votazioni per l'elezione dei componenti dei Consigli di presidenza della Giustizia amministrativa, della Corte dei conti e della Giustizia tributaria, già previste per domani, sono rinviate alla seduta di giovedì 20 aprile.